previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto l988, n. 400,

ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori già prevista per oggi, alle ore 9, è convocata per giovedì 13 maggio 2021, alle ore 9, presso la sede di Palazzo San Macuto.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

desidero rivolgere un commosso pensiero di vicinanza e cordoglio ai familiari, ai colleghi e agli amici del senatore Luciano Modica. Uomo di profonda cultura e brillante intelligenza, Luciano Modica è stato uno dei più autorevoli accademici italiani degli ultimi anni. Siciliano di origini, si era trasferito in Toscana per laurearsi in matematica alla «Scuola normale superiore» di Pisa e intraprendere con passione la carriera universitaria; una carriera di assoluto prestigio, nazionale e internazionale, che lo vide ottenere, a soli trenta anni, la cattedra di ordinario di analisi matematica presso l'Università di Pisa, ateneo di cui solo pochi anni dopo sarebbe diventato giovane e stimato rettore, assumendo nello stesso periodo il delicato ruolo di presidente della Conferenza dei rettori italiani; incarichi che Luciano Modica seppe ricoprire con instancabile dedizione e convinto spirito innovativo. Fu in particolare tra i principali sostenitori degli obiettivi programmatici della Dichiarazione congiunta di Sorbona del 1998 per l'architettura di un sistema superiore d'istruzione europea; un progetto, nel quale - come ebbe a dire in più occasioni - le università italiane avrebbero potuto portare un grande contributo di qualità didattica e scientifica, oltre che storico e culturale. Il suo impegno nella politica attiva era iniziato con la candidatura alle elezioni suppletive svoltesi in Toscana il 27 ottobre 2002 e la successiva elezione al Senato della Repubblica tra le fila dei democratici di sinistra. Nel corso di quella sua unica legislatura come parlamentare, Luciano Modica si è dedicato con grande impegno alle tante questioni legate al mondo dell'istruzione e dell'università. Fu tra i primi a promuovere, con un disegno di legge a sua firma, l'idea di istituire un ente indipendente per la valutazione del sistema universitario e della ricerca; un garante terzo che, senza intaccare l'autonomia costituzionale riconosciuta alle università, potesse comunque contribuire a stimolare un costante miglioramento dell'offerta didattica e responsabilizzare investimenti e strategie di sviluppo degli atenei nazionali: un progetto che Luciano Modica sostenne e contribuì a realizzare nella XV legislatura come Sottosegretario di Stato al Ministero dell'università e della ricerca nel secondo Governo Prodi. Ritiratosi dalla politica attiva nel 2008, era tornato a dedicarsi con inesauribili energie ed entusiasmo allo studio, all'insegnamento e ai tanti progetti rivolti alla cultura, all'università e alla vita e alla vita della città di Pisa, a cui lo univa l'affetto di una vita. Con Luciano Modica perdiamo una persona di straordinario valore umano e culturale, un grande matematico, un saggio interprete delle complesse dinamiche del mondo universitario, un politico equilibrante, dialogante e concreto. In ricordo del senatore Luciano Modica, invito pertanto l'Assemblea

Signor Presidente, alle belle parole che lei ha dedicato nella sua commemorazione a Luciano Modica, vorrei aggiungerne solo qualcun'altra. E partirei con un verbo,

Luciano ha continuato a sostenere il lavoro anche incuriosito dalle modalità con cui ci approcciavamo a provare a sperimentare anche nuovi traguardi e percorsi.

restassero ancorate e in quale modalità si potessero modificare alcuni passaggi, alcuni interventi normativi. Luciano Modica sapeva scrivere le norme

Negli ultimi anni si è dedicato particolarmente a diverse sperimentazioni. Penso a quando ha accolto la sfida, lanciata da noi della Commissione cultura, deputati della scorsa legislatura, sulle lauree abilitanti, che erano una novità e che oggi stanno per vedere il traguardo. Si è dedicato a quella sperimentazione con grande passione, cominciando dal piccolo e da ciò che poteva essere già avanzato. Penso anche alla sua capacità di trasformare in norma trasformare in norma il grande percorso di ascolto che ha poi portato al decreto-legge 13 aprile 2017, n. 59, sulla formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria superiore, ma anche la cosiddetta fase transitoria, curata poi anche dalla ministra Fedeli Fedeli in stretta collaborazione con Manuela Ghizzoni. Per noi che eravamo alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura era comune vederlo insieme al lavoro con la deputata Ghizzoni, nel tentativo di trovare nuove prospettive.

Due giorni fa, proprio con me, aveva avuto modo di raccontare, ancora una volta, il blocco della questione AFAM, a lui molto caro. Lascia un vuoto in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di lavorare insieme con lui. Sappiamo di essere stati davvero dei privilegiati e di aver avuto una grande testimonianza di serietà e professionalità. Anche noi ci uniamo al saluto e alla vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari.

più che mai doverosa l'esigenza di ricordare un collega straordinario che ci ha appena lasciati, Luciano Modica. È una perdita inaspettata che lascia un profondo vuoto non solo nel mondo politico-istituzionale, ma anche in quello accademico, come giustamente lei ha ricordato prima nel suo intervento. Promettente allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa, dopo la laurea in matematica, ha bruciato tutte le tappe della carriera accademica e che, appena trentenne, era già ordinario di analisi matematica all'Università di Pisa,

a disposizione di tutte le istituzioni, come senatore - anche io ho un ricordo personale di quando eravamo eravamo insieme, come ha giustamente ricordato la collega Malpezzi - e poi come Sottosegretario al Ministero dell'università e della ricerca. Lo ricordiamo per l'entusiasmo che lo caratterizzava e che lo ha guidato nella sua attività scientifica, centrata sui numeri e sulle equazioni e che lo ha portato lo ha portato a dare effettivamente un grande contributo politico per molti anni. Uomo di scienza, ma anche delle istituzioni, ha saputo coniugare due mondi apparentemente molto diversi: quello accademico e quello politico. Oggi purtroppo, sia la realtà accademica, sia quella istituzionale si trovano a dover rimpiangere la scomparsa di un intellettuale che ha sempre mostrato il proprio impegno accademico e politico in modo serio e impeccabile e il suo contributo deve per noi rimanere davvero prezioso.

ho conosciuto Luciano Modica all'inizio degli anni Novanta, quando era già presidente della Conferenza dei rettori e quella era una stagione straordinaria per le università italiane, nel senso che c'era un grande fermento. Erano gli anni in cui si stava preparando la legge sull'autonomia universitaria c'era una ricchezza enorme di spunti di riflessione, di creatività nei modelli organizzativi, nella divisione dei *curricula*

che venivano da esperienze importanti di dottorati di ricerca, condotti in collaborazione con strutture internazionali. Luciano Modica, nel suo ruolo specifico di presidente della CRUI, fu il grande regista di quell'epoca: un regista particolarmente attento - per esempio - al tema della valutazione, prima ancora che l'Anvur prendesse forma, a partire da una forte consapevolezza, che era quella della terzietà della struttura che osservava l'università e, osservando l'università, la valutava dall'esterno. Questa ricchezza era preceduta dalla consapevolezza che l'università dovesse essere capace di valutare se stessa. stessa. Ricordo tutto il grande dibattito sugli indicatori di valutazione. L'intelligenza matematica, che chiaramente contraddistingueva il suo modo di affrontare i problemi, lo portava sempre a cercare il corrispettivo quantitativo attraverso la selezione però di un indicatore qualitativo. La gestione che oggi per noi sembra all'ordine del giorno, il grande tema dei *big data*, per lui era già un tema che cercava di far passare in un lungo, lento e profondo lavoro di formazione dei docenti universitari. La grande consapevolezza era che il docente universitario, che normalmente veniva da un'esperienza specifica maturata nel proprio settore scientifico-disciplinare, dovesse imparare a fare il docente in una struttura che era quanto che era quanto di più importante al servizio dell'innovazione e del rinnovamento di un Paese. Prendeva forma con lui quella che oggi è una realtà acquisita, il senso della terza missione dell'università: un'università che non fosse un *hortus conclusus*, rinchiusa in se stessa, ma fosse capace di mettersi in gioco per dialogare, anche con il mondo imprenditoriale. il grande progetto che si chiamava «Più», che significava università e impresa, la collaborazione tra università e impresa e la possibilità dei famosi tirocini aperti, perché gli studenti scendessero in campo e si misurassero con le cose. aveva questa ricchezza, in cui la consapevolezza del rigore del metodo, che gli veniva proprio dalla specificità della sua competenza di matematico, si coniugava con una sensibilità politica e accademica a Furono anni in cui dalla CRUI nacquero tutti i progetti realmente innovativi dell'università. Non nascevano nel Ministero, nel Ministero, oppure nel Parlamento, ma nascevano dalla consapevolezza del ruolo dell'indipendenza dell'intellettuale che esplora il suo sapere, lo rende disponibile e, rendendolo disponibile, in qualche modo si confronta con tutto quello che gli sta intorno. In quegli anni non mi occupavo di politica; mi occupavo di una giovane università che stava nascendo in quel momento.

certamente anche lui ha sofferto del peso di una burocratizzazione di scelte che in qualche modo riusciva forse a fare con maggiore scioltezza nel suo ruolo di presidente della CRUI, a dimostrazione che si può fare una politica di qualità svolgendo diversi tipi di ruoli. Il Parlamento è uno, forse il punto più importante e più qualificante, ma non è l'unico o l'esclusivo. Lo ricordo quindi con grande

il senatore Modica nasce a Catania, come è stato ricordato; poi diventa professore alla Normale di Pisa: brillante carriera accademica da matematico, allievo di De Giorgi. Ha insegnato presso atenei di grande prestigio in tutto il mondo: Parigi, New York University, Edimburgo, Bonn, Minneapolis. La sua carriera politica si avvia nel 2002: nel 2002: eletto durante le elezioni suppletive e successivamente, con Prodi, Sottosegretario al Ministero dell'università e della ricerca. Non conoscevo Luciano Modica ma, per un'incredibile coincidenza, sono amico, stimo una persona che lo conosceva personalmente e lo stimava. Di Luciano Modica oggi, al di là dei meriti strettamente scientifici che riguardano la sua materia, ci restano gli scritti e le riflessioni in ordine alla misurazione delle prestazioni dell'università italiana e della ricerca. Consentitemi di leggere la prefazione di un volume del 2002, a firma a firma appunto di Luciano Modica, in cui scriveva: «L'autonomia dell'università, recentemente completata con la riforma della didattica, pone con forza il sistema universitario di fronte alla sfida della qualità. Gli elementi chiave per vincere questa sfida sono legati alla capacità di tenere costantemente sotto controllo e di misurare quanto viene concretamente realizzato all'interno di ciascuna università; di trasformare queste informazioni in occasioni di apprendimento, di crescita e di miglioramento continuo; di fare di questa stessa capacità di lettura un elemento di trasparenza sempre a disposizione di chi deve scegliere, sia esso studente o decisore politico». Questa mattina ho avuto modo di parlare con l'amico comune che lo conosceva e gli ho chiesto quale fosse la posizione di Luciano oggi di fronte a quegli obiettivi che lui, vent'anni orsono, aveva contribuito a tratteggiare. Mi ha risposto: di grande amarezza, perché negli ultimi anni aveva cercato invano di limitare la deriva burocratica di quel sistema di valutazione. Era molto amareggiato, mi dice l'amico.

atteggiamento critico nei confronti della citata deriva, fosse stato allontanato dalla politica. Mi viene descritto un uomo intellettualmente onesto,

le derive negative che talvolta i sistemi umani assumono, a dispetto delle buone intenzioni. Un uomo così mancherà a tutti perché abbiamo bisogno di uomini intellettualmente onesti. *(Applausi).*

30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena,

il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, reca misure urgenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 e di sostegno ai lavoratori con figli in didattica a distanza o in quarantena. Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di 6 articoli e un allegato. Nell'illustrare il contenuto del decreto-legge, mi soffermerò sulle parti di competenza della 1a Commissione, ovvero sui commi da 1 a 7 dell'articolo 1 e sugli articoli 1-*bis* e 2-*bis*, questi ultimi inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. L'articolo 1, ai commi da 1 a 7, reca alcune misure che hanno in gran parte già esplicato i loro effetti. È stata prevista infatti l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso fra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, volto a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia. In particolare si è stabilita l'applicazione alle Regioni e Province autonome in zona gialla delle misure previste per quelle situate in zona arancione e, per i giorni di festività pasquali del 3, 4 e 5 aprile, l'applicazione su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, delle misure previste per la zona rossa. Sono state quindi disposte le sanzioni applicabili alla violazione delle prescrizioni previste. Inoltre, è prevista e disciplinata una comunicazione quotidiana da parte delle Regioni e delle Province autonome al Ministero della salute del numero dei tamponi eseguiti sul proprio territorio. L'articolo 1-*bis* dispone che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone, ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati o gli imputati, siano consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando i medesimi colloqui siano necessari per salvaguardare la salute fisica e psichica delle stesse persone detenute o internate. L'articolo 2-*bis*, infine, stabilisce che le disposizioni del decreto-legge in esame siano applicabili anche nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. I lavori delle Commissioni congiunte 1a e 11a si sono conclusi senza apportare modifiche al testo approvato in prima lettura presso la Camera dei deputati. Sono stati invece approvati diversi ordine del giorno, fra cui ritengo opportuno menzionare la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1-*bis*.0.1, concernente disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali e *hospice*,

ospedaliera e di ricerca medica applicata Mater Olbia. In particolare, il comma 7-*bis* esclude per il periodo 2021-2026 i posti letto accreditati per tale struttura dal computo relativo al rapporto tra il il numero di posti-letto accreditati a carico del Servizio sanitario regionale e il numero degli abitanti. Si ricorda che la norma generale richiede, al riguardo, che il rapporto non superi il valore di 3,7 posti-letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti-letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie. Il comma 7-*bis* prevede, inoltre, che la Regione Sardegna assicuri, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera, il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati al lordo dei posti-letto accreditati nella struttura in esame. Il comma 7-*ter* estende agli anni 2024-2026 la disciplina transitoria di deroga per la Regione Sardegna, con esclusivo riferimento alla suddetta struttura ospedaliera, al limite vigente della spesa per la remunerazione da parte del Servizio sanitario regionale delle prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. In base alla norma finora vigente, la deroga trova applicazione per gli anni 2019-2023. Il comma 7-*quater* consente che la Regione Sardegna riconosca per un biennio all'ospedale in oggetto i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura. La copertura dei maggiori oneri per la finanza pubblica conseguenti all'eventuale riconoscimento dei costi, ai sensi del presente comma, è assicurata dalla Regione Sardegna. Il comma 7-*quinquies* prevede che il Ministero della salute e la Regione Sardegna assicurino il monitoraggio relativamente alle attività assistenziali poste in essere con la struttura Mater Olbia, alla qualità dell'offerta clinica e alla piena integrazione dell'ospedale in oggetto con la rete sanitaria pubblica, al recupero rispetto ai precedenti flussi di mobilità sanitaria al di fuori della Regione, ai flussi di salute, ai flussi di mobilità sanitaria attiva conseguita. Il comma prevede, inoltre, che il Ministero della salute trasmetta annualmente alla Regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere una relazione sul monitoraggio così effettuato. Riguardo all'articolo 2 si rileva, in primo luogo, che esso prevede per il periodo 13 marzo-30 giugno 2021 la possibilità per i lavoratori dipendenti, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli, di ricorrere al lavoro agile o, in casi più circoscritti e a condizioni che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ad un congedo straordinario con indennità. In particolare, le fattispecie relative al lavoro agile e al congedo straordinario concernono - in alternativa

o di quarantena disposta a seguito di contatto. Si prescinde dall'età del figlio e si consente il cumulo del diritto al lavoro agile tra i due genitori, qualora le fattispecie suddette riguardino figli in condizioni di disabilità accertata o di disturbi specifici dell'apprendimento o di bisogni educativi speciali, nonché per il caso in cui i figli rientranti nelle suddette condizioni frequentino centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per il congedo si prescinde dall'età del figlio e dal requisito della convivenza, qualora le fattispecie summenzionate riguardino figli in condizioni di disabilità grave. Con riferimento ai figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, si prevede, sempre al 30 giugno 2021, il diritto per uno dei due genitori ad un congedo privo di indennità, qualora ricorrano le fattispecie suddette relative al lavoro agile per i figli infrasedicenni. Tutti i diritti summenzionati sono esclusi qualora l'altro genitore non svolga attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, ad eccezione di quelle fattispecie di diritto al lavoro agile che prescindono - come detto - dall'età del figlio. Riguardo, più in particolare, al congedo con indennità, si rileva che quest'ultima è riconosciuta dall'INPS, ovvero dall'amministrazione pubblica datrice di lavoro e che essa è pari al 50 per cento della retribuzione che sarebbe spettata con il riconoscimento ai fini previdenziali della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione. retribuzione. La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali. Di conseguenza, si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. L'importo di tale base di calcolo non comprende il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi, mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore. L'articolo 2 in esame prevede altresì, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e i lavoratori dipendenti del settore sanitario, la possibilità di fruire, entro il 30 giugno 2021, e in alternativa al lavoro agile e ai congedi summenzionati con indennità o senza, della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *babysitting* o di servizi integrativi per l'infanzia per l'infanzia per un figlio convivente minore di anni quattordici, per i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione da Covid-19 o da quarantena disposta a seguito di contatto. Il *bonus* è riconosciuto nella misura massima di 100 euro settimanali. I benefici del congedo con indennità e del *bonus* suddetto sono riconosciuti dall'INPS nel rispetto di un limite complessivo di 299,3 milioni di euro per il 2021. La possibilità di convertire il congedo parentale eventualmente fruito nel periodo dal 1° gennaio al 13 marzo 2021 nel congedo con indennità summenzionata è disciplinata dal comma 4. Il presente articolo 2 reca altre due disposizioni in materia di lavoro agile. Con una norma generale a regime, relativa alla cosiddetta disconnessione del lavoratore, si sancisce il diritto

concordati. L'esercizio del diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. Resta ferma per il pubblico impiego la disciplina del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, l'estensione ai dipendenti pubblici e l'introduzione della fattispecie dei figli con bisogni educativi speciali nella disciplina vigente che, fino al 30 giugno 2021, attribuisce il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave. Il diritto è subordinato, ferma restando la nuova norma più specifica, di cui al comma 1-*bis* del presente articolo 2. Si rileva inoltre che il comma 9 del presente articolo 2 prevede una specifica autorizzazione di spesa, pari a 10,2 milioni di euro per il 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche che usufruisca dei benefici di cui al presente articolo 2. L'articolo 3 reca le norme di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente decreto-legge. Ad esse si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota del ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato il 20 gennaio 2021 e l'impiego delle maggiori entrate conseguenti al suddetto incremento della spesa per il personale delle istituzioni scolastiche, nonché mediante la riduzione per il 2021 di due accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativo agli oneri finanziari derivanti dai provvedimenti legislativi di parte corrente, che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Tale riduzione concerne, nella misura di 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, nella misura di 4 milioni, quello relativo al Ministero della salute. Il complesso degli oneri finanziari derivanti dal presente decreto-legge, costituiti da quelli stabiliti dall'articolo 2 e dall'incremento, in conseguenza del suddetto ricorso all'indebitamento, dell'ammontare degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico, è riportato per i singoli anni nella linea del comma 2.

a discutere in Aula riguarda una soluzione per la vita di tutti i giorni, in un contesto in cui soprattutto

Le soluzioni che vengono proposte sono il congedo parentale o il *bonus babysitting*:

nonostante l'impianto e l'intento siano indiscutibilmente positivi. Il decreto-legge in discussione stabilisce che lo *smart working* di uno dei due genitori sia incompatibile con la richiesta di congedo dell'altro. Con questo impianto sostanzialmente affermiamo che il telelavoro può essere considerato come un modo per conciliare vita privata e impegni professionali: questo - lo sappiamo benissimo - è un falso, è un falso, in quanto il telelavoro, lo *smart working*, è un lavoro a tutti gli effetti. Andiamo nel concreto e immaginiamo un contesto familiare in cui un bambino di otto anni venga posto in quarantena dalla scuola in quanto uno dei compagni è stato dichiarato positivo al Covid; in questo caso, capite bene che ci sarà la necessità di ricorrere alla DAD. Ma come faranno

che di fatto diventa quasi secondaria nell'efficacia lavorativa e nella gestione della famiglia. Dobbiamo però tenere conto anche di un particolare: lo *smart working*, il telelavoro, probabilmente avrà

è incompatibile con la cura e l'assistenza ai figli *under* quattordici in DAD. Per questo chiaro motivo, deve anche essere possibile fruire del *bonus* *babysitter* anche in caso di *smart working*.

alla didattica a distanza per necessità, né nel caso in cui svolgano la propria attività.

Presidente, signori del Governo, non ho alcuna obiezione da fare sulle misure che sono previste e che oggi discutiamo e approveremo in Aula.

non si fonda e non può vantare, salvo in casi molto particolari, un sostegno in forme di insegnamento innovative tali da poter veramente educare alla conoscenza le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole.

durevolmente una condizione del genere. Quello che serve, al di là di un provvedimento come quello di cui stiamo discutendo stamattina, è la messa in ordine di un sistema che consta oggi (in passato abbiamo visto quante difficoltà abbia avuto a crescere e ad andare in ordine) soprattutto di tre fattori. Il primo è la vaccinazione estesa all'intero mondo scolastico. Il secondo è il luogo dove i focolai si accendono, e ripetutamente, che è tutto il comparto trasportistico. Naturalmente dobbiamo prepararci, sì, per la fine di questo anno scolastico, ma in modo particolare - e cito il terzo caso, cioè la stabilizzazione perlomeno di una parte dei docenti docenti precari - per evitare che l'anno scolastico 2021-2022 possa iniziare con le lacune e con le carenze che ha vissuto l'anno scolastico 2020-2021. Sottolineo questo aspetto perché la scuola né in Italia, né in altre parti del mondo ha mai risposto completamente al criterio dell'uguaglianza dell'educazione; chi proviene da una famiglia migliore è in grado di fornire un servizio di conoscenza migliore alle proprie figlie alle proprie figlie e ai propri figli. Con la DAD questa forbice tende ad allargarsi. Se la DAD

parte di una generazione decisiva a una diseguaglianza acostituzionale e a una ulteriore tra Nord e Sud rispetto a quella esistente, che può accendere un'ulteriore frattura nella storia straordinaria

per il reddito del padre, è nella condizione di godere di una serie di vantaggi che quello del mio più caro amico, per la condizione di disoccupazione del padre, non può assolutamente godere; quello che non si può fare è fissare in norma una disuguaglianza.

la situazione pandemica di straordinaria gravità ci ha portato a vivere e a doverci confrontare con scenari nuovi e inimmaginabili fino a pochi mesi fa.

Credo sia necessario un distinguo: durante la prima ondata pandemica della primavera del 2020 con *lockdown* totale, le scuole non erano ben attrezzate ed erano poco pronte a offrire una didattica a distanza. Contestualmente, buona parte delle attività lavorative era ferma e le famiglie sono state in grado di reggere uno scenario, per quanto difficile e preoccupante, compatibile con la vita quotidiana. Tuttavia, negli ultimi mesi, il quadro è profondamente mutato e, se, da una parte, abbiamo assistito ancora a problemi di organizzazione nel sistema scolastico, dall'altra, abbiamo visto come, giustamente, il mondo lavorativo si sia ben organizzato, offrendo possibilità di lavoro in modalità remota per alcune categorie di lavoratori, mentre altre hanno dovuto riprendere in sicurezza la propria attività dal luogo di lavoro. È noto che questa situazione ha comportato molteplici problemi per diverse famiglie italiane, che non erano in grado di assistere i propri figli a casa.

Tutelare le lavoratrici e i lavoratori è una priorità, unitamente al diritto dei minori di essere accompagnati in questa fase di ripresa che, in alcuni rari casi, prevede ancora la didattica a distanza. Non possiamo però non soffermarci, gentili colleghi, su alcuni limiti emersi da questo strumento, non tanto sugli effetti didattici, che non dobbiamo affrontare oggi in quest'Aula, ma su quelli legati al mondo del lavoro. Molte categorie sono state penalizzate e non sufficientemente sostenute; mi riferisco, in particolar modo, proprio al mondo degli autonomi che oggi, come non mai, paga in modo pesante questa difficile situazione economica. Sono molte infatti le categorie che hanno lamentato difficoltà di gestione tra la propria attività lavorativa e quella familiare, poiché, come noto, non è sempre possibile tramutare le proprie mansioni in attività compatibili con il lavoro in modalità remota. Ecco perché, gentili colleghi, il nostro compito è pensare a loro e trovare strumenti adeguati che possano compensare queste categorie per le difficoltà che hanno dovuto affrontare nei mesi scorsi. Infine, sarà compito della politica iniziare a concentrarsi in modo serio sul tema di come conciliare la didattica a distanza, il lavoro da remoto e le esigenze familiari. Siamo tutti certi che con il piano vaccinale andremo incontro a riaperture certe per il mondo scolastico. Ciononostante, non potremo arrivare impreparati ad affrontare un tema così delicato come questo, che ha conseguenze non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche sociale ed economico. Sono sfide importanti, alle quali però, cari colleghe e colleghi, non possiamo assolutamente sottrarci.

ulteriormente restrittivi che hanno riguardato la fase dal 15 marzo al 6 aprile e le chiusure che si sono protratte fino ai giorni di Pasqua, quando tutta l'Italia fu chiusa all'interno di una grande zona rossa.

perché è chiaro che lo *smart working* non sarà soltanto ricordato come un modello di organizzazione del lavoro di questa fase, ma probabilmente in futuro

e necessariamente ciò comporterà la presenza di strumenti di *welfare* adatti a tale tipo di riorganizzazione del mondo del lavoro. Si tratta quindi di un decreto che guarda anche avanti, che fissa una base di partenza per una nuova idea di lavoro e una nuova idea di *welfare* familiare. Va detto, però, che oggi vediamo questo decreto con occhi diversi, perché non c'è dubbio che quelle restrizioni hanno prodotto risultati, possiamo vedere la luce in fondo al *tunnel*, con un tasso di contagio che è sceso sotto il 4 per cento (anche se è vero che va valutato in base alla quantità di tamponi fatti, ma è un dato

non perché il tasso di contagio dipenda dal Governo Draghi, ma perché c'è tutta una serie di provvedimenti messi in campo che denotano un cambio di passo reale. La campagna di vaccinazione finalmente può essere definita tale. È stata necessaria qualche settimana di rodaggio, ma il commissario Figliuolo, incentivato e spinto dal Governo, e la Protezione civile, guidata da Curcio, hanno segnato un vero e proprio cambio di passo. La scorsa settimana sono stati inoculati 2,77 milioni di vaccini, quindi si è raggiunta quella soglia delle 500.000 vaccinazioni al giorno che saranno ormai un dato stabile, anzi si parla di obiettivi più ambiziosi. È chiaro che tutto questo è arrivato perché c'è stata non una manna dal cielo, ma una vera e propria inversione di tendenza nel modo di gestire la cosa pubblica. il Governo Draghi e il fatto di aver chiesto un cambio di passo al Paese nei mesi passati. Oggi questa nostra rivendicazione assume un carattere ancora più importante, perché c'è qualcuno che vuole quasi far pensare che quel cambio di Governo sia stato frutto di un colpo basso e un complotto. Addirittura, qualcuno pensa che questo cambio di Governo sia stato fatto in un *autogrill*. Bisogna avere l'onestà intellettuale di ammettere

Paese. Anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza non è quello preparato dal Governo Conte, ma è stato cambiato quasi per intero e ciò denota che qualcosa non andava bene in quella fase, anche se qualcuno voleva dipingere le cose in maniera diversa. A nostro avviso, c'è bisogno di riaffermare il fatto che, quando le cose non vanno, non si deve gettare la palla sugli spalti, ma si devono affrontare i problemi e cercare di risolverli nel miglior modo possibile.

dovrebbe discutere così come oggi si parla del Covid). C'è infatti bisogno di riscrivere una coscienza comune nel Paese, quando si parla di questioni così importanti, e non utilizzare gli strumenti della comunicazione per delegittimare e denigrare qualcuno. Credo che questo non possa essere il futuro del Paese, che dev'essere governato, anche con contrasti politici e punti di vista diversi, ma mai perdendo di vista l'obiettivo di consentire consentire a tutti di esprimersi, avere un rispettabilità comune e non denigrare gli avversari politici con *fake news* e invenzioni. Occorre cercare di di costruire insieme provvedimenti che diano al Paese respiro, visto che dovremo rilanciare con determinazione l'economia, dopo aver abbattuto i rischi per la popolazione derivanti dal Covid.

disposizione agli aspetti del provvedimento che riguardano gli interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza e in quarantena.

a Pentecoste. Per quanto riguarda l'aspetto della tutela dei lavoratori, crediamo che il Governo abbia perso un'occasione, dimostrandosi

Il Governo perde l'occasione di dare una risposta concreta a milioni di italiani,

che il sistema individuato per i congedi parentali e per il *bonus babysitter* non è parametrato sulle reali esigenze delle famiglie; anzi, mette in grossa difficoltà soprattutto i ceti più deboli, con stipendi più bassi e quindi anche con minore capacità

Camera, sia qui al Senato - rappresenta un fatto dirimente, perché gli aiuti sono insufficienti per tutti, ma per alcuni le misure sono ancora più discriminanti.

la continuazione di determinate attività, nel loro caso della scuola, e non si vedono riconoscere neanche la possibilità di accedere al *bonus babysitter*.

spesso accade - un vuoto impegno che poi non troverà conferma nel prossimo decreto sostegni, con il nuovo scostamento di bilancio. Il personale ATA merita attenzione, come ci è stato segnalato da tantissimi soggetti di questo mondo e dal sindacato Feder.ATA, che ringrazio per il confronto che ha avuto con la nostra parte politica e che abbiamo interpretato, perché nessun italiano dev'essere lasciato indietro. Dimostratelo concretamente: saremo pronti a darvene merito, come lo siamo sempre a dare contributi nell'interesse non del Governo, ma della Nazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, già superato nell'articolo 1, che si riferisce ad un intervallo temporale che va da metà marzo agli inizi del mese di aprile, prevede misure di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Ci dà l'opportunità quindi di focalizzare la nostra attenzione su un tema centrale nella vita del nostro Paese e dei cittadini: la scuola. L'introduzione della didattica a distanza e l'interruzione alternata della frequenza scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado hanno rappresentato fenomeni di assoluta novità, dei quali bisognerà valutare nel tempo i costi sociali. È innegabile che la didattica a distanza non possa essere equiparata a quella in presenza, da ogni punto di vista. I ragazzi fortunati che hanno potuto seguire le lezioni *online* da marzo 2020, senza problemi di connessione o altri inconvenienti, hanno comunque pagato il prezzo di una solitudine forzata, anomala e innaturale. La scuola, come sappiamo tutti, ha pagato uno dei costi più alti della pandemia, vittima della disorganizzazione del sistema dei trasporti locali nel nostro Paese, nostro Paese, la cui inefficienza - non è un mistero - ha rappresentato un ostacolo che ha precluso una riapertura in sicurezza. Neanche con le risorse aggiuntive trasmesse dallo Stato agli enti territoriali si è riusciti a ovviare in breve tempo a problemi strutturali e atavici. Il contesto pandemico, dunque, influendo in modo imprevedibile sull'equilibrio psicologico di molti studenti, ha causato un aumento diffuso di ansia, timori e paure. La mancanza di interazione con il resto della classe e il senso di solitudine causato dall'obbligatorietà del rigore della didattica a distanza rappresentano elementi con cui dovremo fare i conti anche nel prossimo futuro. Nel decreto-legge sostegni parte delle risorse stanziate con l'aumento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sarà rivolta a specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza pedagogica e psicologica. Fare un uso sapiente delle risorse è indispensabile, in primo luogo negli ambienti socio-economici più periferici, arretrati e marginalizzati, dove le famiglie, magari già gravate dalle pesanti ripercussioni economiche, non possono permettersi spese aggiuntive per i figli. In questo contesto pandemico estremamente delicato per l'intero sistema scolastico, gli studenti e le studentesse più fragili, già affetti da forme di disabilità, hanno sofferto ancora di più. Su questo punto vorrei fare una particolare riflessione. Nel decreto-legge di cui stiamo discutendo sono state inserite misure a favore del ricorso al lavoro agile per i genitori nei casi di sospensione delle attività didattiche ed educative dei figli. Certamente, soprattutto nei territori del nostro Paese che hanno più sofferto la chiusura dei plessi scolastici, questa norma, in vigore dalla metà del mese di marzo, può rivelarsi utile per i lavoratori dipendenti. Tale beneficio si estende anche ad entrambi i genitori che hanno figli con disabilità accertata ai sensi della legge 104, del 1992 con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, quindi rappresenta una certa innovazione positiva nel testo del decreto-legge. Tuttavia, allargando per un attimo i nostri parametri di riferimento sulla situazione emergenziale vissuta dagli studenti e dalle studentesse con disabilità, purtroppo, torneranno presto al pettine i nodi irrisolti per lungo tempo. La carenza di insegnanti di sostegno specializzati nei ruoli della docenza rappresenta un *vulnus* cui si sarebbe dovuto far fronte da tempo in maniera più incisiva, così come il raggiungimento dell'accordo in Conferenza unificata che sarebbe dovuto avvenire oltre un anno fa, come previsto nel decreto cosiddetto sulla configurazione dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione. In conclusione, sono queste le figure - l'insegnante di sostegno e l'assistente all'autonomia e alla comunicazione che si occupano ogni giorno degli studenti con disabilità, anche durante la pandemia e con tutte le difficoltà aggiuntive del caso. Se, come affermato dal ministro Bianchi, la didattica a distanza non va vista come ripiego *pro tempore* cosa che giustificherebbe il ricorso emergenziale al lavoro agile - ma come un percorso di integrazione e arricchimento per costruire una scuola nuova, allora ci spieghi il Ministro quale sia la via da seguire per costruire questa nuova scuola. La scuola nuova che vogliamo per i nostri figli non può più permettersi di affidare l'istruzione e l'educazione di ragazzi e ragazze con disabilità a personale non in possesso di specializzazione. Quest'argomento, purtroppo, non sembra essere all'ordine del giorno del questo Governo in carica, e se dunque, almeno per il momento, l'obiettivo di terminare l'anno scolastico in presenza, scongiurando il ricorso alla didattica a distanza, pare essere centrato, non si ha ancora alcuna certezza sul prossimo futuro e su come si intendano affrontare tutte le criticità ampliate dalla pandemia.

scandire tre punti su questo decreto-legge che ci apprestiamo a votare tra pochi minuti. Il primo, com'è stato già segnalato da diversi colleghi, è che ci apprestiamo a votare un qualcosa di già superato.

che, nel momento dell'emergenza, in cui il problema si pone, rendano abbastanza chiaro, in anticipo, cosa le famiglie possono e devono fare per essere attentamente e intelligentemente vicine alle esigenze dei figli e, nello stesso tempo, cosa i genitori o comunque le persone possono e devono fare rispetto al loro lavoro, per riuscire a mantenere insieme la loro responsabilità professionale e di servizio alla comunità e le circostanze e le modalità concrete in cui questo si può realizzare.

in queste circostanze e in queste condizioni. Qualunque sia l'emergenza che le scatena, i genitori devono sapere di poter contare su questo tipo di misure di attenzione e i ragazzi devono sapere di essere tutali da queste misure.

non ho mai visto emergere una proposta molto semplice, lineare e chiara. Perché i nostri docenti di sostegno non riescono a fare propria questa esigenza del docente a domicilio? Ciò non vuol dire

approfondimento delle responsabilità da parte di chi governa tali processi per essere vicini a queste persone. Credo che su tutto questo abbiamo bisogno di fare una riflessione di sistema e di struttura che metta in mano alla scuola, alle famiglie e alle aziende qualcosa di più che non una normativa che ogni tre settimane, come ci avevano abituato i famosi precedenti DPCM, a tambur battente cambia le carte in regola.

è un aspetto molto particolare, che è stato inserito nei commi aggiuntivi all'articolo 1. 1. Mi riferisco a un grande ospedale nato in Sardegna e che va sotto il nome di Mater Olbia. È interessante il fatto che questo grande ospedale appena nato abbia nella sua dizione la parola *mater* sostenere la relazione di cura che evidentemente può e deve mantenere nei confronti dei pazienti. Mi sembra anche un omaggio alla maternità

e nel contesto sociale si nota una specie di pregiudizio nei confronti di tutto ciò che non è interamente, completamente ed esaustivamente statale, come se ciò che viene dal privato vada guardato con diffidenza.

dell'offerta di un servizio di eccellenza sia stata inserita la possibilità di rivisitare alcune norme, avendo presente e centrale il bisogno dei pazienti.

Ci auguriamo tutti che sia veramente un'esperienza positiva, che aiuti l'isola a fare un salto di qualità anche nella sanità che offre.

inviando un abbraccio virtuale, il mio, il nostro come Gruppo della Lega, ma credo quello di tutti noi, alla signora Emma Marrazzo, mamma di Luana D'Orazio, la ragazza che ha perso la vita a Prato. La signora Emma ha lanciato un appello affinché tragedie come quella avvenuta lunedì scorso non si ripetano. Di questa donna mi ha colpito anche la preoccupazione verso la titolare dell'azienda presso la quale la figlia ha perso la vita. In quest'Aula, che rappresenta il popolo italiano e i lavoratori, ripeto con forza quanto espresso ieri in Commissione assieme al senatore Alessandro Ruotolo, ci tengo a dirlo, che ha sollevato il problema,

è ancora ferma. Lo dobbiamo a tutti lavoratori e, soprattutto, a questa ragazza, a suo figlio e a sua mamma, che ha dimostrato un coraggio non comune, lanciando con lucidità un appello a tutti noi. Non si può morire nel 2021 sul posto di lavoro. Chi va al lavoro deve tornare a casa, riabbracciare i propri familiari, i propri cari e non essere pianto. Chiedo quindi un impegno anche alla Presidenza, venga istituita, a prescindere dagli interessi di Presidenza o Vice Presidenza dei partiti. Si tratta di una Commissione importantissima: dobbiamo dare un segnale ai lavoratori italiani. Venendo al decreto al nostro esame, com'è stato detto, è passato: siamo in ritardo anche nell'approvazione, come troppo spesso è avvenuto in quest'Aula. Lo dico con un velo di critica, perché dobbiamo essere veloci per difendere i nostri dobbiamo essere rapidi nel porre rimedio ad alcune esigenze. Si tratta di un decreto contenente alcune misure un ampio ricorso al lavoro in modalità agile per chi ha figli in età scolare, previsione che forse abbiamo sottovalutato, perché abbiamo bisogno anche di socializzazione, e non solo di lavoro inteso come guadagno: non c'è solo l'aspetto economico, ma anche l'aspetto sociale, tant'è vero che abbiamo approvato il *bonus* per servizi di *babysitting* rivolti a genitori lavoratori che non possono svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile e che quindi abbiamo tutelato. Potevamo magari andare oltre i 100 euro settimanali, ma purtroppo la situazione è questa e la pandemia e le problematiche che stiamo vivendo ci hanno imposto questa piccola cifra. Bisogna però tutelare le lavoratrici, le mamme e i papà, affinché vivano con serenità il rapporto familiare con i loro figli, perché è importante: non possiamo pensare solamente all'aspetto economico, perché c'è anche questo profilo. Lo ripeto, perché è importante: c'è anche il livello sociale, la socializzazione fra le persone, il vivere insieme, perché il lavoro è anche libertà di comunicazione, non soltanto uno sterile messaggino, una *e-mail*, un'indicazione lavorativa, ma andiamo oltre: il lavoro è libertà.

per far sì che le persone abbiano tempo libero per vivere i propri rapporti, altrimenti creiamo una società sterile ed eterogenea, perdendo quei valori che hanno reso finora fondamentale la coesione sociale, ossia la famiglia intesa come ente produttivo, sia sotto l'aspetto economico, ma anche sotto quello culturale e di coesione di una Nazione. Per questo, aprendo una parentesi, non molleremo sul concetto di famiglia, perché la coesione nazionale si basa sulla famiglia naturale.

Spero quanto prima di tornare alla normalità, con persone che abbiano la possibilità di tornare sul posto di lavoro, perché bisogna anche dire che ci sono degli effetti collaterali. Con parole semplici, porto un esempio personale, quello della struttura operativa dell'aeroporto, dove intorno

dà le linee guida per lo *smart working* e il lavoro agile, ma non entra nel merito. Per questo a mio avviso dobbiamo scrivere - azzardo questo termine - lo statuto dei lavoratori del digitale,

nel 2023 è riscrivere le regole del lavoro, ma anche della tutela dei lavoratori e delle aziende, perché ad oggi il lavoro agile è lasciato all'interpretazione e alla discrezionalità sia del datore di lavoro che del dipendente,

a tutti i cittadini che hanno fiducia nelle istituzioni democratiche.

per unirci al dolore della famiglia di Luana D'Orazio, una giovane lavoratrice mancata tragicamente mentre lavorava,

Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, oggi in quest'Aula discutiamo un decreto-legge in parte superato, ma credo sia significativo sottolineare, anche *a posteriori*, l'importanza di aver preso misure apparentemente più restrittive del necessario; all'applicazione di misure della cosiddetta zona arancione anche nelle Regioni che avrebbero dovuto essere in zona gialla e, nei giorni delle festività pasquali, all'applicazione di misure da zona rossa su tutto il territorio nazionale. contagio stanno calando anche grazie a queste restrizioni, che ci hanno quindi consentito di poter procedere alle graduali riaperture a partire dal 26 aprile. Da febbraio dello scorso anno ad oggi abbiamo imparato molte cose su questo virus, ma credo che la cosa più importante da tenere a mente sia che non possiamo abbassare la guardia finché non avremo messo in sicurezza almeno la parte più fragile e più a rischio della popolazione. Il calo dei morti giornalieri ci dice che stiamo andando nella direzione giusta, ma sono ancora troppi (ieri sono quindi continuiamo a rispettare le regole: indossiamo le mascherine, manteniamo il distanziamento e igienizziamo frequentemente le mani. Le vaccinazioni stanno procedendo speditamente e, grazie alle consegne finalmente regolari, abbiamo raggiunto la quota di 500.000 somministrazioni al giorno, che ci permetteranno presto di procedere alla vaccinazione di tutti coloro che vorranno farlo. Inoltre, l'EMA sta già esaminando la richiesta di Pfizer di autorizzare la somministrazione per gli adolescenti tra i dodici e i sedici anni, così entro l'autunno potremo proteggere anche i nostri ragazzi in vista del rientro a scuola. Insomma, stiamo andando nella direzione giusta, ma dobbiamo farlo con attenzione e prudenza, perché il nostro primo imperativo dev'essere sempre la tutela della salute. In questo provvedimento ci sono anche altre norme in materia di salute: ci sono, ad esempio, misure volte a garantire l'operabilità del nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata Mater Olbia in Sardegna. Non è un mistero cosa pensiamo del finanziamento indiscriminato alla sanità privata ma, nel momento in cui la struttura esiste ed è stato previsto dalla Regione un sostegno per agevolarne l'avvio e la piena operatività, sarebbe da irresponsabili non consentirlo. I cittadini della meravigliosa Sardegna hanno il diritto - come d'altronde ovunque - di potersi curare nel migliore dei modi nella loro Regione, senza viaggi della speranza verso il continente. Questo dovrebbe consentirlo la sanità pubblica, ma sappiamo bene - l'abbiamo detto tante volte in quest'Aula - come questa sia stata saccheggiata negli anni passati. Abbiamo finalmente invertito la rotta del finanziamento del Sistema sanitario nazionale, ma ci vorrà del tempo per vederne gli effetti. Nel frattempo speriamo tutti che il grande supporto a questa struttura possa colmare velocemente questa carenza e offrire ai cittadini sardi le prestazioni di eccellenza che meritano sul loro territorio, perché quello che manca sono appunto le prestazioni di alto livello e non certo un centro privato convenzionato che offra le prestazioni di livello medio e basso che sono già in grado di garantire le strutture pubbliche esistenti. Infine, nel provvedimento ci sono i permessi parentali retribuiti per i lavoratori in tutti quei casi in cui i figli sotto i quattordici anni non possano andare a scuola o frequentare i servizi educativi. Era inoltre previsto il bonus *babysitter* per i lavoratori autonomi; i colleghi deputati hanno esteso - doverosamente, direi - questa possibilità ai lavoratori del settore sanitario e del comparto sicurezza pubblica e difesa, che purtroppo inizialmente erano stati esclusi.

Ormai da un anno continuiamo a dire che i professionisti e gli operatori sanitari in genere sono gli eroi di questa emergenza; e allora non dobbiamo e non possiamo dimenticarli proprio nel momento in cui approviamo misure a sostegno dei lavoratori. Non possiamo dimenticare chi, fin dal primo giorno, ha pagato un prezzo altissimo per assisterci e curarci. A tutti loro va la nostra gratitudine e aggiungo che possono essere sicuri che continueranno a essere al centro della nostra attenzione e della nostra azione legislativa.

ha sentito una stringente necessità di migliorare le condizioni di vita di tutti i cittadini, oramai stremati economicamente e psicologicamente da questa pandemia. Quando giunge un decreto-legge, ogni parlamentare, spesso incalzato dalle evidenti necessità delle numerose categorie che sono in manifesta difficoltà, vorrebbe presentare emendamenti, alle volte anche non in linea con gli obiettivi dei provvedimenti, per rispondere alle grida di dolore che ci arrivano dalle varie parti del Paese.

Se la Lega sostiene questo Governo, è per amore dell'Italia e degli italiani e per rispetto di quel voto popolare che nelle passate tornate elettorali le ha dato consensi e fiducia. In nome di quella fiducia che il popolo ci ha accordato, noi siamo qui per fare gli interessi degli italiani e gli interessi dell'Italia, in un momento in cui la nostra Nazione non può permettersi di perdere più tempo, perché il tempo per fare qualcosa di concreto è stato perso tra i vari DPCM; a causa di questi ritardi ora noi dobbiamo correre. Vorremmo e dovremmo fare sicuramente di più, molto di più. Penso a tutte le categorie che hanno bisogno di aiuti concreti; anche io avrei potuto ricordare tutte le categorie e presentare dozzine di emendamenti, ma stiamo convertendo un decreto-legge e dubito che la sede per farlo sia il disegno di legge di conversione, anche se siamo abituati spesso a inserirvi di tutto. Dobbiamo tuttavia attenerci all'obbligo di omogeneità del decreto-legge e del disegno di legge di conversione. È quell'obbligo che ci ha rammentato la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, ritenendo *tout court* illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo di omogeneità, un vincolo che la Corte ritiene implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione. Sicuramente ci batteremo affinché tutte le categorie e tutte le famiglie italiane possano ricominciare a vedere un futuro. Ci batteremo affinché i nostri figli possano in futuro frequentare in presenza le nostre scuole, perché lo possano fare in ambienti dignitosi e degni di questo nome. Ci batteremo per tutti i lavoratori, per i nostri anziani, per le persone fragili. Ci batteremo perché nessuno resti indietro e lo faremo con proposte concrete e specifiche.

dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 2-*bis*.1 e 2-*bis.*0.1.

ordini del giorno

depositato per porre in evidenza il grande tema della riapertura delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA), delle case di riposo. Noi chiediamo che venga fatto tutto il possibile per attuare questa riapertura in tempi rapidissimi

preso atto dell'impegno assunto dal Governo in Commissione circa il fatto di intervenire rapidamente con uno dei prossimi provvedimenti, senza attendere

Per quanto riguarda l'emendamento 1.6, noi proponiamo di spostare il coprifuoco almeno alle ore 24 per le zone gialle e bianche. bianche. Come tutti sappiamo, il coprifuoco è una misura di dubbia legittimità costituzionale, anzi secondo noi è assolutamente incostituzionale e viola il preciso dettato della nostra Costituzione,

e soprattutto del fatto che oggi ormai, a maggio, il sole tramonta alle 20,30, c'è luce fino alle 21,30 e non ha alcun senso costringere la gente in casa, dove semmai il contagio si amplifica, mentre all'aperto, come tutti noi sappiamo, il contagio rappresenta soltanto lo 0,1 per cento

non rinviare a chissà quando questa doverosa misura, ma di adottarla oggi e immediatamente. Si tratta di una proposta di buonsenso, non chiediamo nemmeno, come sarebbe giusto, di abolire totalmente il coprifuoco, chiediamo soltanto di estenderlo alle ore 24. alle ore 24. Ai colleghi senatori dico che chi ha il coraggio di assumersi questa responsabilità oggi lo può fare votando a favore del nostro emendamento, che è un emendamento di buonsenso e propositivo.

ora il senatore Balboni.

nelle richieste al Governo di modificare l'attuale situazione. Il nostro sarà un voto di astensione solo perché c'è un ordine del giorno G1.1, approvato in Commissione, a

voluto anch'io ricordare l'ordine del giorno G1.1, che è stato accolto dal Governo in Commissione poche ore fa e quindi ha già dato una soluzione fattiva e concreta alla problematica giustamente posta anche dai colleghi dell'opposizione. Metto l'Assemblea di fronte all'ipotesi di un rischio che potremmo correre: tutti sappiamo che il decreto è in scadenza e c'è il rischio concreto che con l'approvazione di qualche emendamento si vada a far decadere il decreto, facendo quindi perdere tutti i bonus *baby-sitting*, con tutta una serie di conseguenze negative che potrebbero occorrere. Credo che l'approvazione dell'ordine del giorno in Commissione un viatico ampiamente sufficiente per permettere al Governo già nei prossimi giorni di risolvere la questione del coprifuoco.

il fatto che il *virus* va scemando anche in funzione della stagionalità del ceppo virale a cui appartiene, si debba dare un segnale di ritorno alla normalità, di fine di questa emergenza,

impegna il Governo: nel mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese

esprimo parere favorevole a condizione che alla fine siano aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto delle funzioni di programmazione regionale».

Bisognerebbe verificare - come abbiamo fatto noi - il danno alla psiche dei ragazzi che la pandemia sta comportando e agire di conseguenza.

Siamo consapevoli che il ruolo di opposizione, anche patriottico come il nostro, è duro perché si scontra con la volontà di respingere le proposte di buon senso solo perché vengono dall'opposizione. E non salva la coscienza qualche astensione, anzi la peggiora, perché se ci si astiene su una proposta dell'opposizione vuol dire che si è convinti che è una buona proposta ma, siccome viene dall'opposizione, non la si può votare. *(Applausi).* Vincete, allora, contro i nostri emendamenti ma - lo dico senza riferimento ad alcun collega di questa Assemblea - si tratta di vittoria di Pirro, e si sa che Pirro era una persona non intelligente, che non aveva capito che vincere battaglie misere significasse perdere la guerra. Non vorremmo che perdessimo la guerra contro il buon senso. Presidente, condividiamo lo spirito di questo emendamento e abbiamo cercato questa mattina in Commissione di provocare un cambio di atteggiamento. apprezzate le circostanze, il decreto-legge deve essere convertito entro il 12 maggio per cui non ci sarebbero i tempi per un nuovo passaggio alla Camera dei deputati. Abbiamo cercato di cambiare l'atteggiamento chiedendo alle forze di opposizione di

Fratelli d'Italia non voglia trasformarlo in un ordine del giorno al quale diamo sin da adesso la nostra adesione.

parallelamente, in sede di conversione del decreto-legge sostegni, le Commissioni riunite hanno votato un ordine del giorno, che impegna il Governo rispetto a tutta una serie di misure che fanno fronte al disagio psicologico e che dovranno essere inserite, in accordo col Governo, che ha accolto l'ordine del giorno, nel prossimo decreto-legge sostegni *bis* (o decreto imprese), per renderle immediatamente efficaci.

questa grande ingiustizia. Noi, come Stato, combattiamo l'usura; lo Stato non può diventare un usuraio.

la fascicolazione la fate voi.

Siamo in questa situazione: l'emendamento 2-*bis*.1 è stato dichiarato improponibile. Il senatore Vitali dice che in Commissione è stato votato un ordine del giorno che non è pervenuto però all'Assemblea e alla Presidenza. Ci può dire qual è stato il destino dell'ordine del giorno?

testo. Adesso lo accantonerei un momento per poter proseguire con le votazioni. Se ci fate pervenire rapidamente il testo, vediamo di risolvere il problema.

vorrei raccomandare al Governo la massima attenzione su questa vicenda perché, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021, i Comuni già in difficoltà perché in procedura di riequilibrio accompagnato, per effetto della dichiarazione di illegittimità di due commi dell'articolo 39 dell'ultimo decreto milleproroghe, non saranno in condizione di approvare i bilanci di previsione. Parliamo di oltre 800 enti, tra Comuni e Province, ed è necessario un urgentissimo intervento del Governo per salvaguardare gli enti di prossimità ai cittadini che sono proprio gli enti locali.

Signor Presidente, gentili colleghi, da più di un anno siamo ormai in guerra contro un nemico invisibile, ma oggi, dopo tanta trincea, possiamo guardare con più fiducia al futuro. Il cambio di passo della campagna vaccinale ci sta rendendo orgogliosi delle scelte politiche fatte nei mesi scorsi, che hanno portato alla nascita del governo Draghi e alla nuova gestione del commissario straordinario Figliuolo. Lo scorso 30 aprile sono state effettuate più di 515.000 vaccinazioni, con una media, nei sette giorni, superiore a 340.000 dosi somministrate, per un totale di 21 milioni di somministrazioni. Questi numeri fanno luce nel buio dei mesi scorsi e indicano la strada per uscire dal tunnel, ma soprattutto danno la percezione, ma più che la percezione la certezza, di poter raggiungere l'immunità di gregge entro l'autunno. Dobbiamo dare atto che le nostre intuizioni, le nostre coraggiose scelte politiche, si sono dimostrate corrette e ripagano oggi delle tante orribili parole rivolte verso chi con determinazione si prese la responsabilità di assumere decisioni importanti per il futuro della nostra Italia. Grazie al presidente del Consiglio Mario Draghi, nel nostro Paese si è ricostruito un clima di fiducia, di entusiasmo, di autorevolezza internazionale e di speranza per il futuro. Da tempo, e sempre sulla base di dati scientifici, insistevamo sulla necessità di riaprire in sicurezza ed in particolare di far ripartire la scuola in presenza e le attività all'aperto. Oggi riteniamo che si debba lavorare per un ulteriore passo in avanti, rendendo più agevoli gli spostamenti tra le Regioni promuovendo il *pass* vaccinale sia a livello europeo che a livello mondiale. È importante, importantissimo, tornare a vivere. Se prevarrà la responsabilità e se la campagna vaccinale proseguirà come deve, siamo convinti che verrà meno anche la limitazione delle chiusure serali. Siamo felici che la maggioranza abbia trovato con il Governo l'intesa sul coprifuoco; è giusto che si decida sulla base dell'andamento dei contagi e dell'avanzamento delle vaccinazioni: più ci vacciniamo, meno ci contagiamo, prima riparte il nostro Paese. Altre considerazioni invece meritano i ristoratori che non hanno spazio all'aperto e alcune attività sportive che sono ancora bloccate, ma che nei fatti potrebbero operare ed effettuarsi in sicurezza. Il Covid e le restrizioni hanno fatto emergere nuove esigenze di *welfare* familiare e stabilito un nuovo equilibrio tra la vita privata e il lavoro. La pandemia ha cambiato la percezione in relazione ad alcuni temi quali lo *smart working,* i congedi parentali straordinari e il *bonus baby-sitting.*

per uno stanziamento complessivo di circa 300 milioni di euro. Dopo la pandemia lo *smart working* rientrerà sempre di più tra i servizi di *welfare* aziendale, non solo al fine di conciliare in maniera flessibile tutti i momenti della giornata, ma anche per garantire ai lavoratori una maggiore autonomia temporale nell'espletamento dei propri compiti e delle proprie mansioni. Si parla sempre più di *smart welfare* per definire le nuove esigenze dei lavoratori, con le quali dovremo continuare a confrontarci per offrire soluzioni e adeguato supporto. Proprio domani in quest'Aula si tratterà un altro importante provvedimento a sostegno delle famiglie e delle imprese, che mette molte pezze agli errori fatti nel passato. Oggi, consapevoli di aver lavorato bene per il Paese, Italia Viva esprime convintamente il voto favorevole al decreto-legge in discussione. Le sfide che ci attendono sono comunque tante e molto difficili, ma prima di qualsiasi altra cosa dobbiamo pensare alla ripartenza e dobbiamo ripensare alla crescita, al debito buono del Piano nazionale di ripresa

Signor Presidente, ci accingiamo anche noi a fare il nostro intervento di protesta, posto che, come è noto, anche gli interventi di protesta hanno

a disturbo, evidentemente abbiamo una cultura delle istituzioni un po' criptica, un po' *d'antan*, che ricorda altri periodi, magari forse un po' più bui, del secolo scorso. Chiusa questa mi lasci ringraziare invece il collega De Vecchis, che questa mattina ha riportato nella sede opportuna un dramma accaduto due giorni dopo il 1° maggio: il dramma - che evidentemente i colleghi ricordano - è quello della povera Luana D'Orazio, l'ennesima morte sul lavoro. Non è una morte bianca, com'è volgarmente chiamata, ma una morte drammatica e tragica una notizia che ha rischiato di essere cancellata per via di questa celebrazione del 1° maggio che ha catturato l'attenzione sugli *influencer*, sul loro cappellino e

Grazie al collega De Vecchis

alla conduzione d'Aula che l'ha preceduta, perché chiedere il minuto di silenzio dopo che il collega De Vecchis aveva attenzionato questo tema è stato un passaggio a dir poco trasandato e distratto.

per ammissione di tanti degli intervenuti è una sorta di atto dovuto, che ha visto l'Assemblea del Senato impegnata a ratificare,

anche nella indisponibilità - lo dico ai colleghi che hanno sollecitato questo atteggiamento da parte di Fratelli d'Italia a trasformare i nostri emendamenti in auspici, cioè in ordini del giorno. Ci è stata chiesta questa ulteriore disponibilità su vicende di assoluto buonsenso, su cose che abbiamo illustrato bene in Commissione e che fanno parte del dibattito quotidiano che impegna i nostri concittadini. Per esempio, ne dico una che vado spiegando e dicendo da più di un anno in quest'Aula: fare un numero sufficiente di tamponi e di test per individuare l'infezione da Covid-19 nei famosi Come ho spiegato stamattina in Commissione ai colleghi, esistono ormai anche le canzonette che trattano della necessità di scovare gli asintomatici, ma non esistono i provvedimenti di un Governo e di un Ministro che sembra evidentemente aver paura di trovare i positivi al Covid, ancorché asintomatici o presintomatici, capaci comunque di infettare. Altri emendamenti riguardavano la possibilità delle Regioni di circoscrivere le zone rosse a seconda dell'andamento epidemiologico della curva dei contagi; contagi; altri ancora riguardavano la necessità di riaprire le palestre e le piscine o il coprifuoco. Colleghi, si tratta di misure di assoluto buon senso e non di mera protesta, se avessero trovato spazio almeno nella disponibilità del Governo ad esprimere parere favorevole alla loro trasformazione in ordini del giorno, non avrebbero determinato un disagio così grande, forte, enorme, tale da mettere a repentaglio

come ha detto il collega La Russa nel suo intervento dai banchi dell'emiciclo - è che non riuscite ad avere la forza la forza intellettuale di ammettere che ci può essere qualcosa di concreto e di onesto proposto dall'opposizione. Ebbene, non mi sfugge che questo è un gioco delle parti, che ci può stare in condizioni normali, cioè di normale andamento dello scambio democratico dentro l'Aula del Senato; ma non ci può stare in condizioni speciali come questa. La specialità di queste condizioni è data da un lato da un'emergenza che ci trasciniamo da oltre quindici e che ci richiama tutti a un maggior senso del dovere e dall'altro dal fatto che avete una maggioranza così ampia e ipertrofica che evidentemente, invece di aumentare la funzionalità dell'organo (come avviene per ogni ipertrofia), la limita, la condiziona e ne impedisce il regolare funzionamento. colleghi, l'attività e il lavoro di Fratelli d'Italia si moltiplicheranno per far capire quello che sta accadendo in questo momento assolutamente particolare della politica del nostro Paese. In questo tentativo di spiegare l'inspiegabile e in questo tentativo di riportare alla normalità una condizione del tutto del tutto schizofrenica, c'è anche la vicenda che attiene alla da tutti declamata e da nessuno voluta Commissione di inchiesta

dovuto, un ottemperare a un minimo di presenza su un tema drammatico quale quello dell'emergenza Covid-19. Faccio notare, colleghi, che in tutte le legislature è stata istituita una Commissione di inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, senza considerare la vicenda Covid-19. a oltre quindici mesi dalla proclamazione dello stato d'emergenza, figuriamoci se non sarebbe opportuno che il Parlamento si occupasse di questo banalissimo problema. Peraltro, tutte le Regioni stanno normando commissioni di inchiesta sul Covid-19; in quelle governate dal centrodestra lo propone la sinistra, in quelle governate dal centrosinistra (le poche rimaste) lo propone il centrodestra. Il Parlamento, invece, fa come gli strimpellatori del Titanic: la nave affonda e noi, colleghi, ci giriamo dall'altra parte. Anche su questo Fratelli d'Italia è assolutamente lineare e coerente: c'era un testo

ma questa iniziativa si è persa nel nulla, nelle nebbie, nei meandri di un'attività parlamentare che si ferma a ratificare, che si occupa delle pagliuzze e non si occupa delle travi negli occhi dei parlamentari, dei senatori, di quelli che stanno semplicemente nel mondo, girano per i territori e raccolgono le istanze dei nostri cittadini. questa vicenda ci deve vedere seriamente impegnati a rimettere mano all'andamento della gestione della pandemia e alle enormi sfide affronta il nostro Servizio sanitario. Noi abbiamo depositato nuovamente una proposta di legge a questo riguardo, che tiene conto anche dell'emergenza Covid-19; aspettiamo di capire se voi tutti vi renderete disponibili a ottemperare a un dovere assolutamente

rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame è in continuità con quanto è stato fatto negli ultimi dodici mesi: affronta, cioè, importanti aspetti dell'emergenza in corso e si pone nella prospettiva di una gestione efficace delle ripercussioni dirette e indirette della pandemia. Se da un lato è, infatti, necessario mantenere alta l'attenzione sull'andamento dei contagi, dall'altro è però indispensabile anticipare, per quanto possibile, le difficoltà che si presenteranno domani. In particolare, una volta cessata l'emergenza sanitaria - e ci auguriamo che si arrivi presto all'immunità di gregge - ci sarà un'emergenza sociale, economica e psicologica da affrontare. Secondo i dati Istat di marzo 2021, si sono registrati 900.000 occupati in meno, a prevalenza donne, rispetto allo stesso mese del 2020. I redditi da lavoro per le famiglie sono diminuiti di 90 miliardi di euro e le buste paga scese del 6,9 per cento. La nostra economia è in condizioni di grande sofferenza e la politica deve saper dare risposte rapide, risolutive e con capacità di visione e fiducia nel futuro per tutti. La popolazione è stanca e sempre più provata da oltre un anno di sacrifici. Lo scostamento di bilancio già votato potrà senza dubbio contribuire a sostenere ancora le attività con giusti aiuti economici, anche molto anche molto più consistenti rispetto ai precedenti (ne discuteremo a partire da questo pomeriggio); ma allo stesso tempo è urgente affrontare tutte le criticità strutturali emerse in questi mesi e sciogliere quei nodi, superare quei *gap* strutturali che caratterizzano la nostra economia e la nostra società. Il punto centrale è il lavoro. Bisogna ripartire dal lavoro, dagli investimenti che creano lavoro *(Applausi)* - questo è il punto politico di visione e di necessità del Paese per affrontare davvero e darci tutti insieme la prospettiva della piena e buona occupazione, cominciando a sciogliere una per una le questioni decisive che da tempo attendono una svolta. Occorre investire sull'aumento dell'occupazione femminile e giovanile, occorre superare la storica disparità di tutele tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, rivedere in modo serio e organico gli strumenti di protezione sociale dei lavoratori e delle lavoratrici, anche dando seguito e migliorando la sperimentazione delle misure in favore di professionisti autonomi che abbiamo di recente introdotto. Occorre portare a compimento una riforma organica del fisco lo sottolineo, rivolgendomi in particolare al Governo - a partire dall'assegno unico universale *(Applausi)* per costruire un sistema che favorisca la semplicità del rapporto tra lo Stato, le imprese e le famiglie e che incoraggi la la libera iniziativa, la lealtà e la trasparenza fiscale. Occorre poi guardare con spirito costruttivo alle tante novità che si sono affermate durante l'emergenza, a cominciare dalle modalità di lavoro agile, cercando di sfruttarne al meglio le opportunità e di limitare al massimo il rischio di abusi, di riduzione delle tutele e, soprattutto, evitando di scambiare quella che è una diversa modalità di organizzazione del lavoro, delle imprese e delle città con uno strumento di conciliazione dedicato solo ed esclusivamente alle donne

ulteriormente di lavoro non retribuito il lavoro delle donne. Dobbiamo condividere la genitorialità e dobbiamo affrontare, per tutto questo, tutti gli strumenti che rendono effettiva la parità tra i generi per l'accesso al lavoro e nel posto di lavoro. Per tali ragioni riteniamo che l'emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo rischia - se non stiamo attenti a tali aspetti - di esasperare le insopportabili diseguaglianze diseguaglianze che colpiscono le donne e farci fare pericolosi passi indietro. Una delle risposte che è necessario dare velocemente è relativa al divario retributivo che ancora sfavorisce le lavoratrici del nostro Paese. quindi ai contenuti del provvedimento oggi in esame. Seppure limitati a fronteggiare circostanze contingenti, vanno esattamente nella direzione sperata, quella di offrire maggiori tutele ai lavoratori con figli minori o con disabilità, a prescindere dalla tipologia di lavoro, siano essi dipendenti o autonomi. Ricordo l'introduzione, fino al 30 giugno del 2021, di una serie di misure in favore dei lavoratori con figli per fronteggiare l'evenienza, che con la riapertura delle scuole potrebbe ancora verificarsi, della sospensione delle attività didattiche ed educative in seguito a un contagio o alle misure preventive di quarantena. Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti pubblici e privati con figli minori di sedici anni viene innanzitutto riabilitata la possibilità di ricorrere allo *smart* *working* fino a tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche e in caso di infezione da Covid o di quarantena. Questa possibilità è prevista per ambedue i genitori di figli di qualsiasi età con disabilità accertata con disturbi specifici di apprendimento o anche di alunni con bisogni speciali educativi. Per i lavoratori dipendenti con figli minori di quattordici anni è riconosciuta, sempre nel caso di contagio o quarantena, la possibilità di fruire di un congedo straordinario, per tutto o o parte del periodo di sospensione delle attività del figlio, con il riconoscimento di un'indennità del 50 per cento della retribuzione e il versamento della contribuzione figurativa relativo all'intera Si prevede inoltre la possibilità di convertire i congedi fruiti dal primo gennaio al 13 marzo 2021 in congedi straordinari negli stessi termini appena esposti. Anche l'astensione dal lavoro, in caso di impossibilità di lavoro agile, sarà una delle possibilità riconosciute ai genitori con figli da quattordici a sedici anni, sempre nella circostanza di un figlio obbligato in casa. al nostro esame prevede anche un ritorno del *bonus baby-sitting* fino al 30 giugno per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata, autonomi e - lo sottolineo in modo particolare - per il personale del comparto sicurezza, difesa, polizia locale e soccorso pubblico e, finalmente, si

che il lavoro agile non si trasformi in un rapporto di lavoro *non stop* senza orari e senza alcuna tutela, insomma senza più rispetto per i tempi da dedicare alla famiglia, al riposo, allo svago o al benessere psicofisico. Certo, c'è ancora molto lavoro da fare e ce ne sarà ancora di più nei prossimi mesi. I cittadini e le cittadine hanno bisogno di rassicurazioni, è vero, ma come membri del Partito Democratico riteniamo che il Paese abbia bisogno anche di un deciso cambio di passo: che siano rimessi al centro il lavoro e la crescita

condizione di lavoro e di vita, si riaccende la speranza che molti cittadini, donne, giovani e meno giovani ci stanno chiedendo oggi e volendo partecipare anche loro alla prospettiva di rinascita di un Paese

digitale e ambientale. Per queste ragioni, ma guardando sempre di più al futuro, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Ci sono invece molte questioni assolutamente fondamentali su cui il decreto, in particolare con l'articolo 2, continua a espletare tutti i suoi effetti. Mi riferisco a quelle ricordate anche dalla senatrice Fedeli e che riguardano essenzialmente il lavoro agile per il lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di sedici

del congedo straordinario per i lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di quattordici anni e anche per i genitori di figli con disabilità.

la situazione e che ci dice che è necessario mettere in campo delle politiche strutturali per affrontare questo nodo strutturale. Non ci

un investimento fortissimo nella scuola.

una proroga fino al 2026 per quanto riguarda i posti letto e le retribuzioni anche per l'emergenza. Quindi, delle due l'una: o qualcuno ha intenzione di vivere estati calde

per quanto riguarda la Sardegna e anche in ospedali vicini. Affronto ora un'altra questione: abbiamo esaminato anche oggi una serie di ordini del giorno e si è aperto l'ennesimo dibattito sul coprifuoco e sulle aperture. aperture. Su questa vicenda bisogna chiarirsi una volta per tutte, perché - come vedete - nonostante tutte le polemiche su Conte e gli altri, si procede sempre per decreti e noi siamo chiamati a convertire decreti che

si è assunto un rischio ragionato. Quando si dice "ragionato", significa che bisogna ragionare. Quindi, sappiamo perfettamente che verificheremo i dati. Tutti noi speriamo che ognuno usi prudenza che il principio di precauzione sia applicato, perché l'unica cosa che non possiamo permetterci come Paese è che,

Noi voteremo a favore del disegno di legge in esame, con tutte le osservazioni che abbiamo fatto, e spero anche che una volta per tutte si chiuda la stucchevole discussione sull'ora in più e l'ora in meno, quando sappiamo che tutti insieme dovremo vedere i dati e verificarli. Questo

Signor Presidente, gentili colleghi, ancora una volta si discute di un decreto-legge che a che fare con le restrizioni da pandemia Covid, anche se per la verità apparirebbe meno interessante; lo si nota anche dalla scarsa presenza, purtroppo, di colleghi oggi in Aula, perché è un decreto-legge che riguarda provvedimenti che di fatto sono già decaduti. infatti, a restrizioni che ricordano un periodo che si è concluso già lo scorso 6 aprile.

si è di fatto già avviato un processo di nuova speranza e di fiducia riaprendo in quelle ore. In merito alle chiusure serali c'è ormai una decisione che prevede che sostanzialmente a metà maggio - quindi fra pochi giorni - verificheremo quello che l'andamento della pandemia è fondamentale. Oggi ho qui con me una pagina del «Corriere della Sera» che riporta alcune dichiarazioni del generale Figliuolo, ed è giusto che io lo dica a dimostrazione del fatto che ciò che a noi interessa di più è uscire fuori dalla pandemia. E l'unica soluzione perché questo possa accadere è che il piano nazionale vaccinale funzioni a regola d'arte e vada avanti secondo le aspettative del generale Figliuolo. alcuni dati che fanno il seguito alla notizia di soli tre giorni fa: in Italia l'obiettivo che il Governo Draghi si era posto di giungere almeno a 500.000 vaccinazioni al giorno

registriamo con favore anche nella giornata di oggi - fa il paio con un'altra notizia interessante, cari colleghi. Mi riferisco al fatto che da metà maggio avremo il pass verde che forse piacerà molto alla Lega perché è un colore a loro gradito, ma piace anche a me perché amiamo tutto ciò che è verde. Dico bene, cara Sottosegretario.

"rubato" tutti i turisti *(Applausi)*, e questo non lo possiamo permettere. Abbiamo un'offerta straordinaria e siamo in grado di competere ad alti livelli. Queste sono le questioni fondamentali, insieme alle tante altre che pure sono contenute nel decreto-legge in esame, che riguardano il soppresso limite di età per l'accesso dei genitori di figli con disabilità, in situazioni di gravità accertata, al congedo straordinario; l'accesso al lavoro agile consentito anche ai genitori dei figli minori di anni sedici non conviventi; lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile consentito anche per la sospensione dell'attività educativa oltre che didattica. Sono alcune delle misure contenute in questo decreto-legge che sicuramente

con entusiasmo all'invito del presidente Mattarella a comporre, insieme ad altre formazioni politiche, come la Lega, a noi vicina in coalizione, un Governo di unità nazionale. Quando si è in difficoltà bisogna mettersi insieme, superando anche le tante differenze che c'erano, che ci sono e ci saranno con altre formazioni politiche; e ciò per raggiungere gli obiettivi di cui parlavo poco fa,

Signor Presidente, mi consenta una premessa all'inizio del mio intervento. Poco fa abbiamo ricordato la ragazza toscana, morta sul lavoro. Purtroppo, nelle ultime ore, è arrivata la notizia di un altro fatale incidente, questa volta a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in Lombardia, in circostanze simili. Vorrei associarmi, con tutti i colleghi del Gruppo, al dolore della famiglia, esprimendo le condoglianze sia per la ragazza toscana, sia per l'operaio varesino. tornando all'argomento della nostra discussione, con il voto di oggi concludiamo l'esame, nei due rami del Parlamento, del decreto-legge, che, nell'ormai radicato sistema di monocameralismo alternato,

È senz'altro positivo che le norme Covid vengano ora stabilite con un decreto-legge, norma di rango primario, e non più con i DPCM di Conte e Casalino, ma siamo ancora lontani dal pieno coinvolgimento del Parlamento. Oggettivamente, in questa specifica occasione ciò era difficilmente attuabile, visto che le norme in questione, valide per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile, compresa la Pasqua in zona rossa, di fatto erano già superate addirittura durante l'esame in prima lettura alla Camera Sarebbe quindi stato un mero esercizio accademico andare ad intervenire nel merito, essendo la cosa del tutto inefficace, non essendo noi dotati di una macchina del tempo. Anzi, l'approvazione di qualche emendamento improvvidamente presentato avrebbe magari riclassificato qualche zona rossa in zona gialla e avrebbe magari stabilito che qualche attività a marzo avrebbe potuto aprire. Ma l'emendamento non può far apparire dal nulla i clienti e i conseguenti incassi, riguardanti il mese di marzo. Cari amici di Fratelli d'Italia, l'unico effetto sarebbe stato la perdita dei ristori: oltre il danno, anche la beffa. Questo è l'effetto di un'opposizione fatta per partito preso e non obiettiva. C'è però da prendere atto, con soddisfazione, che la stagione dei divieti totali è terminata. Il terrorismo mediatico di chi vorrebbe vederci tutti rinchiusi eternamente in un *bunker* antiatomico di sovietica memoria è stato surclassato dal pragmatismo del presidente Draghi presidente Draghi *(Applausi)* che, parlando di rischio calcolato, ha dato il via alla stagione delle riaperture. Ciò è stato possibile perché in questo Governo, alle posizioni miranti ad una anacronistica ed eccessiva prudenza, si è contrapposta la voce della Lega e di Matteo Salvini riaperture serali dei ristoranti, anche se per ora solo all'aperto, e la ripresa di alcune categorie di attività sono solo l'inizio. Ora bisogna procedere speditamente e sempre e solo dove i dati scientifici lo consentono. È una condizione che intendiamo ribadire e sottolineare con decisione: sempre e solo dove i dati scientifici lo consentono. procedere a verifiche, con cadenza rapida, e ad ulteriori *step* di apertura. Chiediamo prioritariamente la cessazione o, in subordine, lo slittamento in avanti dell'orario del coprifuoco serale. Per la ristorazione ci sarebbe un duplice vantaggio: sanitario, con la possibilità di diluire le presenze in una fascia oraria più ampia, ed economico perché consentirebbe un duplice turno di clienti. Con l'arrivo della bella stagione e il progredire della campagna vaccinale si deve permettere di tornare a un'attività sociale, anche in fascia serale, che, se svolta all'aperto - come dimostrato da più studi scientifici - non è a discapito del contenimento dei contagi. L'approvazione di poco fa dei nostri ordini del giorno sul coprifuoco e sulle riaperture è un impegno netto che il Governo si è assunto. C'è un'altra tematica che, come Gruppo Lega, vogliamo portare all'attenzione dell'Assemblea e lo facciamo ancor più convintamente dopo che la Camera ha inserito nel provvedimento l'articolo 1-*bis*, che permette facilitazioni per le visite ai carcerati.

Decine e decine di migliaia di persone da più di un anno non possono vedere i loro cari. Ora sono tutti vaccinati e non c'è motivo di tenere in vita questa limitazione. Facciamo loro più danno a privarli di un abbraccio e dell'affetto di uno o più familiari. Se vogliamo procedere con cautela, si dia almeno rapida attuazione alla nostra proposta di consentire quantomeno l'accesso alle RSA a chi è in possesso della certificazione verde. l'abbiamo istituita, usiamola per qualcosa di sicuramente utile che permetterebbe anche di vedere con maggior simpatia ciò che al momento è percepito come un ulteriore fardello burocratico, limitante e negativo. Permettiamo da subito - mi appello al Governo - a chi è vaccinato, guarito dal Covid o ha un tampone negativo di entrare nelle RSA e riabbracciare nonni, nonne, padri e madri. Nelle ultime ore sui *media* e, forse in una sede ancor più importante, stamattina in Commissione il Governo si è espresso in tal senso e, quindi, siamo ampiamente fiduciosi. Con questo auspicio, con lo spirito di responsabilità che contraddistingue il mio Gruppo, dando fiducia alle scelte del presidente Draghi, che ha dimostrato di saper ascoltare, oltre che di saper fare, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier.

Governo, onorevoli colleghe e colleghi, per la difficile battaglia contro il Covid-19, anche ora che la campagna vaccinale sta finalmente decollando e prendendo il giusto andamento sia in termini di programmazione che di organizzazione, oltre che di maggior partecipazione, raggiungendo anche le 500.000 somministrazioni al giorno, restano di importanza fondamentale l'ampia e convinta adesione dei cittadini; il loro spirito di solidarietà e di appartenenza alla comunità e il convincimento in ognuno di noi che i propri comportamenti corretti influenzano più o meno direttamente lo stato di salute degli altri. I maggiori ostacoli riscontrati fino ad oggi nella programmazione della lotta al Covid-19 sono da ricondurre al realizzare il giusto equilibrio tra i diversi provvedimenti sanitari ed economici che necessariamente coinvolgono e si ripercuotono sul nostro vivere sociale. Tali misure ovviamente devono essere capaci - da un lato - di limitare e contrastare la circolazione e la diffusione del virus e delle sue emergenti varianti, abbassando così la curva dei contagi dall'altro - le stesse non devono sconvolgere ancor di più di quanto accaduto finora la struttura economica del nostro Paese, il suo tessuto sociale, con il coinvolgimento degli stessi difficili equilibri familiari. Non è un problema di sproporzionata rigidità o di eccessiva cautela. Il tutto scaturisce dalla necessità ovvia di procedere con la dovuta e massima attenzione. Siamo di fronte a un virus estremamente aggressivo e diffusivo. Lo dimostrano i milioni di vittime nel mondo e i dati dei contagi nella loro fredda e asettica rilevazione. Credo che tutti quelli che all'inizio affermavano incautamente che quanto stava accadendo nella fase iniziale della pandemia era gonfiato quasi ad arte o straordinariamente eccessivo, per cui le chiusure, le restrizioni e i *lockdown* adottati erano sproporzionati rispetto alla reale gravità e che, al contrario, occorreva aprire tutto, alla fine si sono dovuti completamente ricredere, dovendo obiettivamente riconoscere che la prudenza e le misure di sicurezza adottate fossero indispensabili, magari da discutere nella loro complessità o da smussare in alcuni passaggi, ma necessarie e non differibili. In questo difficile e purtroppo lungo percorso tutte le misure e i provvedimenti - secondo me - sono stati e dovranno essere ispirati e guidati da un criterio di gradualità e di progressività. Non si tratta di essere rigoristi o aperturisti. Non vi possono essere due fazioni di fronte ad un unico nemico, il virus. Si tratta di essere semplicemente equilibrati nelle decisioni e commisurati nelle scelte. Occorre procedere in questo difficile passaggio che ci dovrà portare fuori dal tunnel della crisi pandemica, affidandosi sempre alla scienza, alle misure suggerite dagli studiosi e ai dati oggettivi, relativi agli indici di contagio dei vari territori e ai consequenziali tassi di occupazione delle terapie intensive. Tutte queste informazioni, insieme ad altre, fotografano perfettamente e oggettivamente la realtà epidemiologica e devono guidare le consequenziali scelte politiche. Indubbiamente occorre anche coraggio nelle decisioni e nelle scelte, che non deve significare però spregiudicatezza. Al contrario, vi devono essere la giusta consapevolezza, logicità e consequenzialità nei provvedimenti adottati. Ragionare con razionalità e obiettività, senza lasciarsi andare a entusiasmi sproporzionati, ma adottando scelte logiche, chiare e assolutamente proporzionate alla gravità del momento: solo in questo modo si potranno evitare scelte di cui poi pentirsi e da cui potrebbero scaturire dannose retromarce. Non si possono fare voli pindarici o cavalcare l'onda del populismo o semplicemente contrastare, gridare allo scandalo e affermare inopinatamente che tutto è sbagliato e tutto è da rifare, un comportamento che non tiene assolutamente conto dell'oggettività relativa alla situazione epidemiologica. I dati dei contagi sono cifre incontestabili di cui prendere atto e su cui riflettere. Non esiste una regola del «tutto è giusto» o del «tutto è sbagliato». Esiste solo il buon senso del confronto responsabile e della condivisione delle scelte. Il principio che deve guidare i nostri comportamenti e le nostre scelte deve essere unico e ben chiaro. La salute del singolo cittadino va messa al primo posto. Uno sforzo comune, al di là delle diverse posizioni politiche, è indispensabile e deve essere fatto, così come altrettanto impegno e sacrificio vengano chiesti a tutta la collettività. Tutti noi lo dobbiamo attuare nel doveroso e sentito rispetto delle tante sofferenze e delle decine di migliaia di vittime che il Covid-19 ha provocato e continua a mietere. Il Governo Conte aveva tracciato un percorso, pur tra le tante difficoltà e le molteplici e complesse problematiche che ne hanno reso difficile il cammino: ostacoli questi ultimi da ricondurre, non solo alla pandemia, ma spesso a veti incrociati e contrapposti, fatti aprioristicamente, nella ricerca risultata vana di visibilità e di consensi o anche nel tentativo, non riuscito, di scalfire la popolarità e il consenso di chi quel Governo lo guidava nel momento più drammatico e critico della pandemia per il nostro Paese. Le misure adottate in questo come in altri provvedimenti, come d'altronde lo stesso PNRR, vanno nella direzione di quel percorso già intrapreso, pur con le ovvie variazioni e gli aggiustamenti necessari, riconducibili alle modificate situazioni epidemiologiche generali e alla disponibilità di dosi vaccinali sempre maggiori. tutto ciò rappresenta un implicito ed indiretto riconoscimento della bontà del lavoro svolto da Giuseppe Conte e dal Governo da lui presieduto Il MoVimento 5 Stelle ha dato e continua a dare la sua fiducia ad un Governo che si muova in tale direzione e sia impegnato costantemente a proporre misure e provvedimenti che tutelino prima di tutto la salute dei cittadini, in particolare dei soggetti più fragili e delle categorie più a rischio. Al tempo stesso, tali misure costituiscono un sostegno concreto alle persone più in difficoltà e una tutela per chi ogni giorno vive realmente sulla propria pelle le drammatiche conseguenze della crisi. Il MoVimento 5 Stelle c'è sempre, ogni giorno e per tutti. È presente e lavora nell'interesse del Paese. Annuncio pertanto il voto favorevole del

del Sars-Cov-2 cominciamo a conoscere molte cose, sia perché ci sono molti studi scientifici, sia perché comincia a esserci il dato dell'esperienza sappiamo che, come molti *virus* respiratori, come i coronavirus più frequenti, anche questo è un virus stagionale; lo abbiamo visto la scorsa primavera e la scorsa estate quando i contagi si sono affievoliti

ma portando il Paese fuori dall'emergenza. In particolare, critico fortemente la mancata approvazione di quegli emendamenti che avrebbero consentito di riaprire già da oggi le attività di palestre, piscine, scuole di danza, insomma di tutto ciò che si poteva fare sempre nelle zone gialle e nel rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria. Allo stesso modo critico fortemente la mancata occasione di estendere la possibilità di tenere aperti i locali e di poter circolare liberamente anche dopo le ore 22, ovviamente sempre nelle zone gialle, e quindi dove non ci siano *cluster* o particolari situazioni di contagio alto. Questa opportunità non è stata colta e il Parlamento in realtà non è stato messo nella condizione di discutere pienamente di queste misure, anche misure, anche perché noi ci troviamo a dover convertire decreti-legge che hanno già esplicato la loro efficacia nel momento in cui noi li convertiamo. Torniamo alla normalità, con attenzione ma senza fare terrorismo mediatico.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, siamo alla conclusione della prima lettura in Senato del decreto-legge sostegni; un percorso che ha unito i Gruppi parlamentari nell'intento di dare risposte efficaci al Paese, ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori, agli studenti, su cui la crisi si sta accanendo sempre più. Ringrazio il Governo, i ministri Franco e D'Incà, il vice ministro Castelli qui presente, i sottosegretari Bini e Durigon, i Presidenti delle Commissioni finanze e bilancio, i Capigruppo e i commissari tutti, i funzionari e gli Uffici, nonché il correlatore, senatore Manca, per il lavoro svolto nelle Commissioni e per lo spirito di vera collaborazione che ha caratterizzato l'attività pur nel distinguo delle diverse sensibilità dei vari Gruppi parlamentari. Permettetemi anche di ringraziare l'opposizione, che ha contribuito alla conclusione positiva dell'esame di questo provvedimento. Il Parlamento ha finalmente riacquistato un ruolo centrale nel processo legislativo, perché la sua azione, in occasione di questo provvedimento, è stata senza dubbio incisiva, sia per la significativa attività emendativa al testo del disegno di legge, sia per aver impegnato il Governo, attraverso ordini del giorno votati in Commissione, ad affrontare altri temi richiesti dal Parlamento nel decreto sostegni- Il percorso nelle Commissioni per la conversione del decreto-legge ha visto i Gruppi parlamentari individuare proposte emendative che responsabilmente possano dare risposte efficaci a chi sta fuori dal Palazzo e che in questi mesi ha visto e purtroppo continua a vedere morire i propri cari, la propria attività, il proprio lavoro; svanire i propri sogni; perdere gli anni più spensierati della giovinezza e i periodi fondamentali di attività didattica, determinanti per la crescita personale e per il futuro di un'intera generazione. Pertanto, a livello parlamentare sono stati individuati alcuni grandi temi, su cui si è trovata convergenza senza spezzettare le risorse disponibili in tanti rivoli impercettibili e perciò inefficaci. temi di grande portata, a partire dal sostegno alle imprese relativamente ai costi fissi, che le stesse devono comunque sostenere anche se impossibilitate ad operare pienamente.

la sospensione al 100 per cento del canone RAI per tutto il 2021 per le attività cui è stato imposto di non lavorare, incluse quelle inerenti al terzo settore; le agevolazioni fiscali per i locatori che nel 2020 hanno subito morosità, oltre all'istituzione di fondi da dedicare al completamento dei cicli di dottorandi e provvedimenti a favore dei bus turistici, delle *startup*, delle emittenti locali. Altre misure sono a sostegno delle fragilità, come l'istituzione del fondo per i genitori separati o a sostegno del turismo, come il fondo dedicato alle terme e quello per la valorizzazione delle nostre città d'arte e dei nostri borghi. Importante è il fondo dedicato al *welfare* aziendale e alle società sportive dilettantistiche,

anche se sarebbe stato qui necessario un intervento più radicale con una vera e propria proroga per differire una norma che non è conciliabile con il periodo pandemico che stiamo vivendo e la conseguente crisi economica. Da segnalare inoltre sono il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela della salute per i professionisti. Nel piano vaccinale è stata inserita, inoltre, la priorità di accesso ai vaccini per i malati oncologici in *follow-up* e la possibilità di effettuare i vaccini alle infermiere volontarie della Croce Rossa. Insomma, si tratta di una serie di misure che a livello parlamentare hanno completato il decreto, ma che saranno ancora più efficaci in combinazione con gli altri impegni richiesti al Governo per il provvedimento sostegni-*bis* attraverso un ulteriore intervento sui costi fissi come la riduzione della Tassa e la proroga e l'ampliamento del credito di imposta per le locazioni ad uso non abitativo; le iniezioni di liquidità alle imprese attraverso nuovi fondi di garanzia dello Stato e una moratoria per i mutui esistenti; preziose risorse per la ripartenza. richiesti inoltre una maggiore attenzione ai lavoratori stagionali e un incremento di 100 milioni per il settore della montagna. Tutto questo completa il decreto che già di per sé si distingue dai precedenti ristori per la *ratio* con cui è stato concepito attraverso l'allargamento della platea dei destinatari dei contributi a fondo perduto e l'eliminazione delle cruciali criticità derivanti dall'utilizzo dei codici Ateco, pur nell'invariata disponibilità delle risorse - ricordo 32 miliardi - votate con lo scostamento dello scorso gennaio, risorse con cui si sono dovuti affrontare più temi. Il provvedimento si compone di cinque titoli. Il titolo I è dedicato al sostegno alle imprese e all'economia con gli articoli che includono i contributi a fondo perduto per le imprese, con una copertura di copertura di 11,15 miliardi di euro; il sostegno per il settore della montagna; l'implementazione del fondo per i lavoratori autonomi e professionisti di un 1,5 miliardi di euro; e ancora l'intervento riservato agli adempimenti fiscali attraverso la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente di riscossione e l'introduzione dell'annullamento dei debiti a residuo fino a 5.000 euro dei singoli carichi relativamente al periodo dal primo gennaio 2000 al 31 settembre 2010 per i redditi non superiori a 30.000. Successivamente si fa riferimento all'incremento di 420 milioni per il fondo dedicato alle utenze elettriche e alla tariffa del canone RAI che - come sopra ho evidenziato - l'attività emendativa ha voluto completare. Il titolo II prevede disposizioni in materia di lavoro, essenzialmente incrementando la cassa integrazione, prevedendo indennità per i lavoratori stagionali del turismo e dello sport, senza tralasciare le misure a sostegno delle fragilità, esoneri contributivi per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Il titolo III prevede misure in materia di salute e sicurezza, stanziando 2,8 miliardi di euro destinati ai vaccini e farmaci per la cura del Covid e 51,6 milioni per i Covid hotel. Il titolo IV concerne gli enti territoriali con interventi da 1,5 miliardi in favore dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province; il rimborso delle spese sanitarie delle Regioni per le emergenze per l'anno 2020; il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle entrate non percepite tramite l'imposta di soggiorno. Rientrano in questo titolo anche il fondo istituito presso per il MEF per il sostegno alle attività economiche delle Regioni colpite dall'emergenza e il fondo di 800 milioni per supportare il trasporto pubblico locale nel 2021. Al titolo V invece appartengono le altre disposizioni urgenti, le misure per favorire le attività didattiche e per il recupero delle competenze degli studenti, anche per quanto riguarda il sostegno delle attività scolastiche in forma digitale per le Regioni del Mezzogiorno, le misure a sostegno delle università e della formazione artistica e di ricerca e, ancora, la tutela delle persone con disabilità, misure per la funzionalità delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, delle Capitanerie di porto, delle Forze armate, la proroga dell'operazione «Strade sicure», che con l'attività emendativa è stata sostenuta con 10 milioni di euro, e tutte le misure per il sistema delle fiere, delle filiere produttive, per la cultura e per la Protezione civile. Ora il decreto sostegni è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 marzo, tardi rispetto ai precedenti ristori votati prima di Natale e rispetto all'acuirsi della crisi, ma nei primissimi mesi di quest'anno si sono verificati gli avvenimenti che tutti conosciamo: la crisi e la caduta del Governo Conte II e l'istituzione del Governo Draghi. Già dai primi provvedimenti, compreso il presente, si è segnato un cambio di passo che è stato confermato con l'elaborazione finale del PNRR, piano fondamentale per la ripartenza e il futuro del sistema Paese, reso significativo dall'integrazione di contenuti della nuova stesura e poi inviato a Bruxelles nei termini previsti. Ecco i passi in avanti che si auspicavano con la nascita di questo nuovo Governo di unità nazionale e di salute pubblica, Governo che ora, con le vaccinazioni, le riaperture graduali e il miglioramento progressivo dei provvedimenti, grazie a un Parlamento partecipativo, darà un impulso efficace a quanti stanno chiedendo da mesi e mesi aiuti concreti. È chiaro che sarebbe stato auspicabile realizzare ulteriori provvedimenti a sostegno del Paese e che si può e si deve fare meglio, ma è altrettanto evidente che solo il riavvio verso una nuova, ma piena normalità favorirà la ripresa della nostra economia e soprattutto della nostra vita.

lavorato con intensità e con grande spirito di collaborazione. Voglio partire da questo primo ragionamento, condividendo tutta la relazione che la correlatrice senatrice Toffanin ha appena svolto, Toffanin ha appena svolto, perché, a mio avviso, è significativo dell'identità che abbiamo voluto dare a tale percorso di collaborazione che ritengo essere una bella pagina di collaborazione proficua e positiva tra Parlamento e Governo. C'è stata infatti una grande collaborazione della struttura tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze, che non va mai dimenticata, a cominciare dal capo di Gabinetto, dottor Chiné, ma in rappresentanza di tutte le diverse articolazioni di un Dipartimento delle finanze assai importante, perché vi si riscontrano i criteri fondamentali propri anche dei principi costituzionali: l'imparzialità e la professionalità sono elementi decisivi per salvaguardare il futuro del Paese ed elementi di terzietà che credo siano da ribadire di fronte ad ogni provvedimento, perché vi è stato un percorso molto lungo e complesso. e complesso. Da diversi mesi la crisi pandemica ci costringe a leggi di bilancio praticamente sotto falso nome, nel senso che sono decreti che in realtà hanno nella complessità di una legge di bilancio l'elemento fondamentale da cui dobbiamo partire. Questa collaborazione, quindi, è stata vera e reale ci ha consentito anche di costruire grande convergenza nelle forze politiche di maggioranza che sostengono questo Governo e soprattutto di lavorare anche con le opposizioni, di lavorare anche con le opposizioni, pur nella distinzione dei ruoli, all'interno di una leale collaborazione, che ha determinato alcune intese che hanno insieme consentito la conclusione di un percorso non banale, né scontato, ma molto complesso, che ovviamente il decreto-legge in sé racchiudeva.

reale. La crisi pandemica ha richiesto tante misure di limitazione di molte piccole attività ed era giusto rispondere a questa domanda di aiuto, che rischiava di essere anche una contrapposizione tra Istituzioni e piccole realtà che avrebbe potuto produrre conflitto

per una prima importante riduzione dei costi fissi delle imprese corrisponda al primo dovere che abbiamo, ossia intervenire per dare una risposta all'abbattimento dei costi fissi e ricostruire una leale collaborazione tra lo Stato e le piccole attività economiche che sono state fortemente colpite

di centinaia di migliaia di partite IVA e attività alle quali abbiamo tolto un'insopportabile tassa che andava azzerata per tutto il 2021 come elemento e contributo decisivo di alleanza, ripartenza e ripresa insieme delle attività.

Queste due misure, che insieme all'esenzione dal pagamento del canone RAI valgono 430 milioni di euro, sono condivise - hanno dato dignità alla leale collaborazione tra il Parlamento e le realtà economiche più fragili e deboli, coinvolte in una crisi pandemica molto complessa. È un primo segnale - non l'ultimo

una forma di assistenzialismo inutile, ma rappresentano la precondizione per evitare che una crisi pandemica si trasformi in un gigantesco conflitto sociale. Saranno poi necessarie le riforme e dovremo riformare quest'istituto, ma la crisi pandemica ci ha dimostrato che il primo obiettivo che il Governo ha introdotto - - quello di non lasciare sole le persone - era una decisione fondamentale per tutelare la coesione sociale del Paese ed evitare un conflitto che avrebbe potuto produrre danni seri anche al futuro e alla ripartenza dell'economia e della società.

al lavoro e all'impresa, proprio per evitare un conflitto sociale, è stata, a mio avviso, una scelta giusta, perché qui stiamo operando sui 32 miliardi di scostamento autorizzati (si tratta del penultimo scostamento, perché l'ultimo votato votato in quest'Aula sarà utilizzato dal decreto sostegni-*bis*). Tuttavia, queste misure di oltre 200 miliardi portano l'Italia tra i primi Paesi europei, insieme alla Germania, ad aver utilizzato risorse fondamentali per la competitività economica, oltre che per la tenuta della coesione sociale. Avremo avuto limiti, sicuramente, perché una crisi pandemica introduce sforzi inimmaginabili e non prevedibili, ma credo che la strada intrapresa sia stata giusta, coraggiosa e importante e ad essa dobbiamo guardare con grande attenzione e grande senso di responsabilità. Il terzo sostegno riguarda la salute. Abbiamo introdotto in questo decreto-legge tutte le risorse necessarie non solo per acquisire i vaccini, ma per dare velocità al piano di vaccinazione. ma per dare velocità al piano di vaccinazione. Averlo fatto portando le vaccinazioni a circa 500.000 giornaliere ha rappresentato e rappresenta la prima misura economica per ripartire: questa è la questione cruciale. Chiaramente, il decreto ci mette nelle condizioni di disporre di risorse sufficienti per realizzare tale grande, primo e importante obiettivo di questo Governo: velocizzare il piano di vaccinazione è la prima misura economica per uscire dalla crisi pandemica.

Le fragilità sociali abitano nel territorio: aver messo al centro importanti interventi di sostegno agli enti locali e alle Regioni; aver reso più flessibile il debito di una Regione; infine, aver garantito ai Comuni le condizioni fondamentali con risorse aggiuntive per coprire il mancato gettito delle prestazioni che in pandemia non potevano generare entrate, sono state, a mio avviso, scelte fondamentali e decisive per la tenuta di questo Paese. Paese. Questi quattro sostegni ai pilastri più importanti segnano una continuità delle risposte, ma anche una volontà precisa del Governo di dare un'accelerazione importante alla prima misura economica fondamentale, che è la tutela della salute e il piano di vaccinazione.

È una scelta giusta, che ci mette tuttavia anche nelle condizioni di predeterminare un indirizzo fondamentale, che abbiamo condiviso e votato in Commissione, che è quello di dare elementi fondamentali per indirizzare il prossimo decreto. Questo per me ha una valenza politica grande, perché è forse una delle prime volte nelle quali ci sono sintonia, sinergia e allineamento anche rispetto a come il Governo attuerà il prossimo decreto in Consiglio dei ministri. Abbiamo dato un indirizzo preciso su alcune tematiche fondamentali. Le ricordo velocemente per questioni di brevità,

perché lì si rischia di consumare un problema reale. Secondo aspetto fondamentale del prossimo decreto: introdurre misure aggiuntive per i Comuni a sostegno delle fragilità. cioè deciso di dire al Governo che è necessario occuparsi immediatamente delle fragilità che abitano nel territorio, perché la crisi pandemica lascia ancora nel territorio i problemi delle fragilità sociali. Occorre un fondo ulteriore per aggiungere risorse al sistema delle autonomie locali per contrastare le fragilità. Ancora, abbiamo introdotto una prima misura per abbattere i costi fissi, ce ne sono altre, a cominciare dall'eliminazione della Tari per chi ovviamente è stato chiuso e deve continuare a ridurre costi fissi per le attività economiche.

la necessità del confronto. Il disagio psicologico tra i minori è una questione cruciale per il futuro di questo Paese. Si è detto al Governo che serve un fondo straordinario per aggiungere risorse ai consultori, per allargare un diritto, quello di contrastare il disagio psicologico dei giovani. sarà un tema del prossimo provvedimento, ed è un'iniziativa importante che abbiamo intrapreso e che, insieme alle altre misure, determina un intervento ulteriore nel mondo del lavoro per i lavoratori cosiddetti stagionali, quelli più fragili. Il mondo dello spettacolo e della cultura contempla aree di precarietà che esistevano già prima della crisi pandemica: aver chiesto al Governo di utilizzare il prossimo provvedimento per risolvere questi limiti è un altro elemento fondamentale della conversione

va attribuito a una grande responsabilità di coesione della maggioranza che, pur di fronte a identità differenti, ha preso tra le mani quella più importante, che è l'interesse nazionale, nazionale, che credo rappresenti una pagina positiva del lavoro parlamentare e del ruolo del Parlamento anche in relazione al Governo.

abbiamo affrontato e commentato il decreto-legge sostegni - primo provvedimento di aiuto alle imprese e all'economia nazionale del nuovo Governo Draghi - con la stessa obiettività e con la stessa onestà intellettuale con le quali ci siamo approcciati ai provvedimenti del precedente Governo Conte

approdato in Aula. Il DEF, infatti, evidenzia una revisione al ribasso delle stime di crescita per l'anno in corso rispetto a quanto previsto dal documento programmatico di bilancio dello scorso ottobre: si passa da una crescita programmatica del 6 per cento a una del 4,5, motivata dal DEF come conseguenza della ripresa dei contagi e delle nuove restrizioni. Una situazione, quindi, certamente figlia della pandemia, ma anche di una gestione poco attenta all'equilibrio tra le esigenze sanitarie e quelle economiche, che ha costretto di fatto molte imprese e molti settori a rimanere chiusi senza precise evidenze scientifiche che ne attestassero la pericolosità. Di conseguenza, è lo Stato a cercare di porre rimedio attraverso l'intervento pubblico, che si è rivelato, ahimè, poco efficace. Sempre con onestà intellettuale, in tema di indennizzi alle imprese, o ristori, che dir si voglia, abbiamo accolto con soddisfazione trattandosi peraltro di due modifiche chieste a gran voce da Fratelli d'Italia, proposte ripetutamente nei nostri emendamenti ai provvedimenti del Governo Conte - l'estensione dei contributi a fondo perduto alla platea dei professionisti e il superamento della logica fredda dei codici Ateco. Ateco. Ancora, con la stessa lucidità intellettuale, non possiamo non ribadire l'inadeguatezza dell'ammontare dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto-legge, a favore soprattutto del mondo produttivo: erano inadeguati i ristori del precedente Governo Conte e lo sono egualmente quelli dell'attuale Governo Draghi, a maggior ragione considerando il perdurare dell'emergenza sanitaria che aumenta sempre di più le difficoltà del mondo produttivo. Parliamo di contributi che, a seconda del volume d'affari, vanno dall'1,7 al 5 per cento del fatturato perso complessivamente nell'intero 2020. Credo che già questo dica tutto e le percentuali si commentano da sole, purtroppo. Si tratta piuttosto di una presa in giro, che non di qualcosa che possa definirsi un contributo: non saprei come altro definire quei 2.500 euro per un commerciante, un artigiano o un ristoratore che nel 2020 hanno subito una perdita 50.000 euro, magari dimezzando il loro fatturato rispetto all'anno precedente. Questo è il caso più favorevole, perché, salendo il volume d'affari, come detto, la quota del contributo diminuisce rispetto alla perdita subita. subita. Purtroppo, sul tema non vediamo sostanziali differenze rispetto ai decreti-legge ristori del Governo Conte; vediamo, anzi, assoluta continuità, e a dirlo sono le cifre, che evidenziano come siano quasi praticamente identici negli importi. Le cifre sono impietose anche sotto l'aspetto del lavoro. Siamo scesi in piazza il 1o maggio, mentre altri ascoltavano concerti o comizi improponibili, da palchi autorevoli.

La CGIA di Mestre ha stimato, per il solo 2020, una perdita di fatturato complessivo, per le imprese italiane, di circa 423 miliardi di euro. A fronte di questo, il Governo Conte ha destinato alle imprese 11,3 miliardi di euro, a titolo di contributi diretti a fondo perduto, pari ad appena il 2,7 per cento del fatturato perso. Il decreto-legge sostegni ha stanziato poco più di 11 miliardi di euro: la cifra è simile, ma la platea è più vasta, comprendendo anche i professionisti ed avendo eliminato ovviamente i codici Ateco. alle precedenti, arriviamo a ristori che coprono il 5,3 per cento del fatturato perso nel solo 2020. Il presidente Draghi ha affermato che il Governo si è mosso nell'ambito dei 32 miliardi di euro di scostamento di bilancio già approvato: si poteva fare di più per le imprese e le partite IVA,

che mettesse a terra manovre diverse, ma non siamo i soli, perché il decreto-legge sostegni è stato addirittura bocciato dalla stessa maggioranza, considerato che sono stati presentati complessivamente oltre 3.000 emendamenti, dei quali meno del 15 per cento erano di Fratelli d'Italia, unica forza all'opposizione: il rimanente 85 per cento erano della maggioranza, che in questo modo sconfessa l'operato stesso del suo Governo. Proprio per questo ci aspettavamo di più, anche dal passaggio nelle Commissioni, in cui abbiamo provato a migliorare il provvedimento, con proposte che andassero nel verso di un intervento per sostenere completamente i settori in crisi e lo abbiamo fatto attraverso emendamenti puntuali. Come abbiamo detto nei mesi scorsi, era necessario in primo luogo intervenire sui costi fissi, che gravano sulle imprese, in quanto la logica del *bonus una tantum* non risolve il problema del mondo produttivo e della continuità imprenditoriale. Se non lo risolveva prima, a maggior ragione non lo fa ora, dopo un anno di chiusure e restrizioni. Abbiamo ribadito per questo la necessità di intervenire a copertura dei costi fissi che gravano su imprese, artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, quali, ad esempio, canoni di locazione, mutui e *leasing* in essere, utenze, imposte e tasse, premi assicurativi, versamenti contributivi, quando indipendenti dal fatturato, come nelle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti. Invece il decreto-legge prevede poco o nulla in tal senso. Qualche piccolo passo avanti è stato fatto con alcuni interventi approvati nelle Commissioni, che hanno previsto ad esempio l'esenzione totale dal pagamento del canone RAI per le strutture ricettive e per i locali di somministrazione o anche la proroga dal 30 giugno al 30 dicembre dell'esenzione della tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Lo stesso vale per l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU per le imprese che nel 2020 hanno subito un calo di fatturato almeno del 30 Si tratta comunque di interventi di portata molto limitata e per l'appunto insufficienti, a maggior ragione se si considera che nel 2020 è terminato per quasi tutti i settori anche il credito d'imposta del 60 per cento sui canoni di locazione degli immobili utilizzati nell'attività di impresa. Per gli altri settori è terminato il 31 dicembre 2020, dopo averne beneficiato per i mesi da marzo a giugno e da ottobre a dicembre. Fratelli dall'Italia a tal proposito ha presentato due proposte emendative al decreto-legge, che sono state trasformate, nel corso dell'*iter* in Commissione, in ordini del giorno, che impegnano il Governo a valutare l'opportunità di prevedere ristori commisurati ai costi fissi e l'estensione dei crediti di imposta sulle locazioni. Sempre in tema di locazioni, accogliamo positivamente il fatto che in un emendamento al decreto-legge sia stata prevista la non tassabilità dei canoni di locazione non percepiti dal proprietario dell'immobile locato, come da tempo proposto da Fratelli d'Italia, anche in relazione al decreto-legge sostegni. Positiva è la novità che riguarda i professionisti. Grazie a un emendamento presentato da Fratelli d'Italia, è stata approvata la misura che riconosce il principio del differimento per malattia Covid dei termini relativi agli adempimenti che i professionisti devono rispettare a tutela di questi ultimi e dei loro clienti. tutti, bisogna approvare il disegno di legge di Fratelli d'Italia per estendere i diritti anche a quelle categorie che fino ad oggi si sono sobbarcate il costo delle loro malattie. estendere l'applicazione dei regimi facoltativi della cedolare secca e del canone concordato anche per gli immobili non abitativi, prevedendo la possibilità di optare da parte del proprietario per la stessa tassazione prevista per i canoni di affitto derivanti dagli immobili a uso abitativo. Anche questa è una proposta di Fratelli d'Italia.

Riteniamo necessario tutelare i settori di rilevanza strategica dalle scalate ostili da parte di aziende straniere che potrebbero approfittare della debolezza del tessuto finanziario, economico e sociale del Paese come conseguenza della nuova ondata pandemica. Alla luce anche del recente caso Iveco, abbiamo proposto di estendere al settore automobilistico l'uso dello strumento della *golden power*. Allo stesso tempo, abbiamo proposto di prorogare l'esercizio dei poteri speciali al 31 dicembre 2021 in tutti i settori strategici e, in particolare, quelli finanziari, bancari e assicurativi, dell'agroalimentare e del siderurgico. A questo proposito, balza agli occhi il cortocircuito interno alla maggioranza relativamente all'articolo 37, la cui finalità è intervenire per supportare con una finanza ponte anche le aziende in amministrazione straordinaria e a cui, in realtà, i tempi di approvazione del decreto-legge di fatto impediscono di avere liquidità in tempo breve. Porto un esempio che conosco: la Acc di Trichiana, un'azienda del mio territorio, paga sulla propria pelle la carenza di liquidità. È una diatriba tutta interna alla maggioranza tra chi ne riconosce il progetto come strategico, e quindi meritevole di intervento pubblico, e chi invece crede che a intervenire debbano essere i privati. Peccato che a rimetterci siano i dipendenti, illusi da mesi di promesse non mantenute. Questa è l'unica discontinuità che abbiamo visto sul campo tra il Governo precedente e questo, ma in peggio. per le imprese che hanno subito un calo di fatturato nel 2020 che la variabile passi dal 25 al 33 per cento a seconda del volume d'affari. Sulla scuola, tenendo fede alla nostra linea politica e per dimostrare di essere un'opposizione costruttiva non solamente - come leggiamo oggi da qualche agenzia - una che grida e basta, abbiamo proposto soluzioni per la mobilità straordinaria per l'eliminazione del vincolo quinquennale, il concorso riservato solo per i direttori dei servizi generali amministrativi, l'aumento dell'aliquota per la mobilità interprovinciale, la mobilità straordinaria per i dirigenti scolastici. Da parte nostra, ci sono fatti e non parole in favore del personale della scuola (precari, dirigenti scolastici e personale ATA).

- sono le istituzioni di prossimità ai cittadini e che sono in prima linea nel combattere l'emergenza Covid. Avevamo segnalato per primi che i Comuni non riuscivano ad approvare i bilanci entro il 30 marzo e con un emendamento avevamo già proposto di prorogare il termine al 31 marzo.

all'articolo 4, che definiamo una mezza rottamazione, che non è né carne, né pesce e che serve a poco, se non alle esigenze dell'amministrazione per abbassare il magazzino fiscale. Ai cittadini e alle imprese serve davvero poco, perché è limitato a un importo di 5.000 euro e a coloro che hanno un reddito entro i 30.000 euro lordi l'anno. Si tratta di una misura inutile e ingiusta, perché si rivolge a una fetta di popolazione estremamente limitata e che potrebbe giovare giovare ai cattivi pagatori che lo sono per negligenza e non per errore. Avevamo proposto la sospensione delle cartelle e una maggiore rateizzazione, dando così risposte non solo a qualcuno.

all'emergenza Covid non possono essere perimetrate in gabbie normative, come effettuato dai vecchi decreti. Ci vuole flessibilità. Bisogna concedere alle Regioni che le rendicontazioni vengano considerate come un unico finanziamento e le varie risorse assegnate dai quattro decreti, prescindendo dai limiti finanziari che i vari commi dei singoli articoli prevedono per ciascuna linea di attività. Un'emergenza si affronta con strumenti emergenziali, non con quelli ordinari.

il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi è solamente un piccolo tassello all'interno di un più ampio quadro di aiuti e sostegni che, da un anno a questa parte, Parlamento e Governo stanno mettendo in atto per provare a fornire un supporto concreto a fronte della crisi che sta attraversando il Paese ormai da troppo tempo. Tutti abbiamo la consapevolezza che non si tratta di soluzioni definitive né risolutive, soprattutto per i tanti operatori economici che hanno dovuto ridurre, in maniera talvolta drastica, la loro attività e che, proprio a causa di questa crisi, sono stati costretti a scelte molto difficili e, addirittura, anche alla chiusura delle loro attività. C'è ancora molto da fare ed è per questo che il Governo è al lavoro già da settimane per varare il prossimo decreto sostegni, che sarà approvato a giorni e su cui tutti lavoreremo, per migliorarlo. Oggi, tuttavia, siamo chiamati a discutere e a votare un provvedimento che costituisce un passo importante. Il lavoro fatto dal Parlamento è stato assai significativo ed è andato anche nella direzione giusta. Tanti sono stati gli emendamenti approvati in Commissione e di questo, ovviamente, dobbiamo rendere grazie ai suoi membri che hanno lavorato molto bene e che hanno cercato di raccogliere le istanze di tutte le categorie, o quasi perché qualcuna è sicuramente rimasta fuori. A questo riguardo, non posso non pensare all'incremento del fondo da destinare alle imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea, che erano state escluse dai precedenti provvedimenti; o, ancora, all'esenzione della prima rata IMU per i soggetti che svolgono attività di impresa, di cui ha parlato il relatore poco fa; imprese che producono reddito agrario. Ancora, vi è un importante contributo all'Ospedale pediatrico Bambin Gesù al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19, nonché da quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni ad alta complessità proprio in conseguenza della pandemia. pandemia. Alcuni emendamenti insistono sull'esigenza che probabilmente in questo momento è quella maggiormente sentita, cioè quella di accelerare i vaccini. Noi di Italia Viva, da questo punto di vista, siamo stati i primi a sostenere la necessità di un'accelerazione della campagna vaccinale in questo senso, non possiamo che ringraziare il presidente Draghi, che si è impegnato e continua a impegnarsi in maniera assolutamente fattiva su questo tema. Consentitemi anche un ringraziamento al generale Figliuolo che, fino ad oggi, ha rispettato in maniera assolutamente precisa tutti gli impegni che aveva preso e anche i programmi che si era dato e che sta continuando a darsi. Siamo certi che i risultati non tarderanno a vedersi. In quest'ottica, l'emendamento voluto da Italia Viva introduce la possibilità anche per le strutture alberghiere, che hanno patito moltissimo la crisi, di diventare *hub* vaccinali a disposizione del sistema sanitario italiano, per accelerare il più possibile i tempi e facilitare l'accesso di tutti coloro che ancora si devono sottoporre alla vaccinazione. Grazie all'impegno di Italia Viva è stato approvato anche un importante emendamento, fornisce un aiuto concreto per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo e, in particolare, nel settore della movimentazione dei *container* e nell'attività di trasbordo merci. L'emendamento porta anche la mia firma: l'ho fortemente voluto, anche perché sollecitato da miei corregionali e da colleghi parlamentari alla Camera dei deputati, alla Camera dei deputati, convinto che sia necessario e non più procrastinabile intervenire, dando un ausilio reale ed effettivo agli operatori portuali fortemente colpiti dall'emergenza epidemiologica.

discorso riconosce un'indennità ai lavoratori in esubero dei porti per cui si è realizzata una sensibile diminuzione del traffico rotabile e passeggeri e al contempo permangono stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche delle imprese portuali. La nostra volontà è dunque quella di sostenere fortemente l'occupazione al contempo di evitare gravi pregiudizi all'operatività e all'efficienza portuali.

Con questa misura, quindi, ci occupiamo finalmente di un settore che fino a questo momento sembrava poco considerato, ma che deve tornare a essere centrale anche e soprattutto per i lavoratori impiegati nei porti che hanno vissuto e stanno vivendo in prima persona una crisi dovuta, appunto, all'emergenza pandemica. Mi auguro però - e ci tengo a dirlo - che questo sia solo il primo segnale per la Sardegna in materia di trasporti marittimi; auspico che ci sia una maggiore attenzione di quella manifestata fino ad oggi

testo in discussione costituisce sicuramente una svolta e, come dicevo, sarà seguito a breve da un secondo decreto sostegni. Con esso abbiamo raggiunto alcuni importanti traguardi per dare un effettivo e concreto sostegno a tutti coloro che, a vario titolo e in vario modo, sono stati colpiti da questa crisi, crisi, dando anche un segnale di speranza a tutti quei settori che ancora devono essere coinvolti e ai quali ovviamente assicureremo tutto il nostro impegno per far sentire che non ci siamo dimenticati di loro. Cercheremo invece di far sentire la nostra presenza e di riavviare l'Italia, che di questo ha davvero tanto bisogno. Siamo certi però che con la guida che abbiamo al Governo questi risultati riusciremo a portarli a casa.

vorrei sottoporre alla sua attenzione la valutazione di improponibilità dell'emendamento 39.0.66 (testo 2) per due ragioni: estraneità alla materia e rispetto alla competenza delle Commissioni Quanto all'estraneità alla materia, il decreto-legge contiene disposizioni dirette ad affrontare la crisi economica generata dalla pandemia. Si tratta di misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori; inoltre, più in particolare, non contiene alcun intervento a regime per la materia ambientale. L'emendamento approvato in Commissione modifica il codice dell'ambiente per sottrarre la posidonia spiaggiata alla disciplina dei rifiuti, così da poterla considerare risorsa. È dunque evidente che ci sia estraneità. Aggiungo che il decreto-legge ha come fondamento una situazione emergenziale, che non sussiste invece con riguardo all'emendamento 39.0.66 (testo 2), che ritengo debba essere dichiarato improponibile, pena la violazione dell'articolo 77 della Costituzione, quindi l'approvazione di un provvedimento incostituzionale, con conseguente fondato

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottrarrò pochissimo tempo alla vostra attenzione, anche perché corro il rischio di sembrare ripetitivo. Quando si parla della mancata attenzione nei confronti dello sport, purtroppo bisogna ripetere sempre le stesse cose, ma non importa, perché questa materia merita il rispetto che le si deve. un settore in crisi - lo abbiamo detto più volte - e forse più di tanti altri non è stato attenzionato come avrebbe dovuto.

difficile affermazione sotto il profilo della fattispecie giuridica, ma ciononostante ha avuto riconoscimenti da parte dello Stato, e di questo ovviamente non possiamo che compiacerci. Si sta sempre più affermando, in tutti i provvedimenti che abbiamo esaminato nel corso di quest'anno pandemico (e non sono stati

La battuta che viene sempre più spesso ripetuta in questi contesti è che avremo lavoratori, ma arriveremo al punto che non ci saranno più i datori di lavoro. È un'affermazione importante, che oserei definire drammatica e che si scontra con quello che sta accadendo all'interno del mondo dello sport. Abbiamo cercato di correggere questa impostazione in chiave emendativa; ci abbiamo provato in tutti i modi. Non ci resta che andare a denunciare con chiarezza, con decisione e soprattutto che abbiamo provato a correggere questa impostazione, ma ci è stato detto di no. Allora è giusto che il mondo dello sport sappia a cosa è stato detto di no. Nel decreto-legge sostegni l'unico riferimento al mondo

ci sono stati infatti provvedimenti che riguardavano i possessori di partita IVA e, nel caso specifico, tutte le aziende che si occupano di attività sportive o di gestione di impianti sportivi sono state ricondotte al mondo delle piccole e medie imprese. Quindi c'è stato un richiamo totalmente indiretto. C'è però una grande difficoltà che

tra i requisiti necessari per avere un'agevolazione c'era il possesso della partita IVA. Ebbene, il 90 per cento delle associazioni sportive non è in grado di avere questo requisito, e questo le ha escluse.

Siamo opposizione responsabile e, quando parliamo di responsabilità, sappiamo anche vedere quello che di buono all'interno di un provvedimento è stato fatto, non tanto nella prima stesura, quanto nella fase emendativa. In questa circostanza, abbiamo ritenuto opportuno sottoscrivere due emendamenti della maggioranza, uno del centrodestra, che che ha differito l'entrata in vigore del decreto sul lavoro sportivo al dicembre 2023, e un altro importante, a prima firma del senatore Errani, che ha circoscritto gli effetti della concessione dei *voucher*. Si tratta di un provvedimento importante; mi verrebbe in mente - citando una frase del senatore Agnelli - che solo la sinistra può fare cose di destra. *(Applausi)*. Nel caso specifico, la sinistra si è ricordata dei datori di lavoro, cercando di andare a trovare quell'equilibrio all'interno del decreto tra lavoro e azienda, tra lavoro e impresa. Bene, sono atteggiamenti da opposizione responsabile, che continuerà a segnalare a questo Governo, in termini di vigilanza, cosa dovrà essere fatto, senza trascurare la possibilità di convergere su ciò che è giusto e su ciò...

vorrei provare a soffermarmi sul senso che hanno queste misure,

cioè di coloro che sono inghiottiti già ora nelle sabbie mobili della povertà. Vorrei provare ad avanzare questo ragionamento, anche perché penso che il mio partito, il Partito Democratico, debba essere innanzitutto quello dei non garantiti nella nostra società. Vedete, cari colleghi, la pandemia ha inasprito di molto la contrapposizione,

I settori più colpiti vanno evidenziati, perché non è che la pandemia abbia colpito indistintamente tutti: turismo, tempo libero,

la cui occupazione è crollata con la pandemia, alle famiglie povere con bambini, ai lavoratori giovani e agli immigrati. Di fronte a tutto questo, le Commissioni congiunte finanze e bilancio hanno reso un buon servizio al Paese,

un passo importante verso le piccole imprese più penalizzate dalle chiusure e un motivo di soddisfazione per tutto il nostro Gruppo politico.

Pesco e D'Alfonso, tutti i componenti della maggioranza, la disponibilità attenta e costante del Governo e la posizione non pregiudiziale dell'opposizione.

Un pacchetto ampio, che si collega a quello che verrà nelle prossime settimane, al decreto sostegni-*bis*, che interverrà in maniera ancora più focalizzata sul tema dell'impresa; che si collega anche al piano vaccinale, che sta andando avanti in maniera spedita, e al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è stato appena inviato a Bruxelles. Tutto ciò ci deve far guardare con più fiducia al futuro, senza facili ottimismi, ma con misurata e determinata positività. Parafrasando Churchill, confesso che ci stiamo avviando verso giorni migliori.

la conversione in legge del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, all'attenzione del Senato oggi, rappresenta l'occasione per ribadire la necessità di operare scelte concrete e veloci nell'interesse del Paese, che ha subito ulteriori rallentamenti in termini di crescita e di occupazione a causa della pandemia. Sono stati mesi difficilissimi per le partite IVA e, in particolare, per le piccole imprese impegnate nel turismo, nella ristorazione, nel commercio. Le misure del *lockdown* imposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19 hanno messo in ginocchio tante piccole aziende, alcune delle quali non ce l'hanno fatta a sopportare il carico senza introiti e hanno gettato la spugna e abbassato le saracinesche definitivamente. Il calo dei consumi delle famiglie, la cassa integrazione, lo *smart working* hanno inciso profondamente sui fatturati delle piccole attività, Per questo ho apprezzato che siano stati inseriti dei correttivi: la cancellazione della prima rata IMU per le attività che hanno registrato un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'anno precedente e l'istituzione di un fondo per ristorare i Comuni per i mancati introiti, cosa molto, molto giusta per assicurare i servizi essenziali

chiaramente di una boccata di ossigeno, non della soluzione definitiva al problema, per le imprese impegnate nella somministrazione di cibi e bevande che in questi mesi sono state costrette a lavorare solo con l'asporto (e per molti non è stato neppure possibile). A questo proposito lancio un appello al Governo, per rivedere l'orario di chiusura dei ristoranti e dei bar, per lo meno fino alle 23, tanto per dare tempo agli avventori di consumare una cena in tranquillità e di dare serenità al lavoro di cuochi, camerieri e baristi. Spero presto si possa consumare pasti anche all'interno delle sale, rispettando distanze e misure di prevenzione. Questo chiedono gli addetti ai lavori della ristorazione. Allo stesso modo, spero che si possano rivedere le misure per dare possibilità a tutto il settore *wedding* di ripartire; è un comparto importante, con esso ripartono i fiorai, le aziende che si occupano degli abiti da ricevimento, i fotografi e tutte le aziende del *renting.* Accanto ai provvedimenti approvati, rilevo con molta soddisfazione l'approvazione di due emendamenti che incrementano il fondo previsto rilancio per sostenere il comparto della ceramica artistica e tradizionale, rendendo disponibile una cospicua cifra, pari a 4 milioni di euro, che potrà essere utilizzata dal settore. Mi sento di ringraziare, oltre chiaramente al senatore Manca e alla senatrice Toffanin per il lavoro svolto in Commissione e all'intera Commissione, i senatori Lanza e Collina, che sono i primi firmatari di due emendamenti importanti, uno dei quali porta anche la mia firma, e tutti i componenti dell'intergruppo parlamentare per le città della ceramica artistica e tradizionale, di cui sono lieta di essere La nascita dell'intergruppo, infatti, è stata particolarmente importante; continueremo a lavorare in sinergia e sono certa che riusciremo a portare avanti significativi progetti per supportare il mondo della ceramica e sostenere un comparto fondamentale per tante Regioni italiane, compresa la mia Campania, e per la città d'arte di Cerreto Sannita nella provincia Le botteghe di ceramica sono rimaste completamente chiuse durante il *lockdown*, non hanno potuto lavorare; necessitavano, quindi, di avere attenzione. Spero solo che questi fondi saranno di supporto all'attività primaria dei ceramisti e che non saranno soltanto ristoro, ma offerta di lavoro con delle committenze reali che diano dignità ad un comparto che è vanto del *made in Italy*. Mi auguro altresì che non si farà soltanto promozione, perché in questo modo non sarebbero evidentemente protagonisti gli artigiani, ma si possa fare anche formazione; gli allievi potrebbero andare per esempio nelle botteghe, come attività extracurriculare per imparare quest'arte meravigliosa direttamente ai torni, manipolando argilla. In questo modo si raggiungerebbero due obiettivi: guadagno per i ceramisti e formazione per gli studenti. Ci sono imprese e lavoratori che sono rimasti fuori dal decreto-legge, che pure meritavano di essere sostenuti. Voglio richiamare i fuochisti,

per loro vede tempi lunghi a causa del divieto di assembramento. Presidente, anni di investimenti e sacrifici su professionalità ed attrezzature non possono essere liquidati, anche perché consentono di rinnovare le tradizioni popolari e religiose in tante comunità italiane. Al Governo chiedo di sostenere questi settori messi in ginocchio dalla pandemia,

segnali concreti alle partite IVA. Per queste ragioni esprimo il mio favorevole, anche se rimane sicuramente ancora tanto da fare.

povertà, a favore della salute e della sicurezza, di sostegno ad enti territoriali. Si poteva fare di meglio? Si poteva fare sicuramente di meglio. Si poteva fare di più? È un po' difficile dire se si poteva fare di più. Teniamo conto, onorevoli colleghi, che il nostro debito pubblico ha sfondato i 2.650 miliardi. Noi stiamo impegnando il futuro non più dei nostri figli, ma anche dei nostri nipoti. Stiamo giocando tutto sulla buona spendita del *recovery fund*,

presentati molti emendamenti. Devo dire che il lavoro dei relatori è stato imponente e coadiuvato dalla capacità, dall'impegno e dalla costanza degli uffici. Credo che il Governo abbia dimostrato sensibilità su questi problemi e ritengo non vi sia differenza tra destra, sinistra e centro; quando si parla dei bisogni vivi, della gente che lavora o che non lavora più e che vuole lavorare, dobbiamo essere, siamo stati e saremo sempre tutti insieme. C'è stato l'impegno da parte del Governo di accogliere degli ordini del giorno che rappresenteranno la struttura portante del prossimo decreto-legge sostegni. Stiamo licenziando il primo e già stiamo pensando al secondo. Ciò dà l'idea

quale deve essere il rapporto tra la politica, intesa come Parlamento ed Esecutivo, e la burocrazia ministeriale, cioè con quegli uffici di diretta competenza del Ministero che io chiamerò burocrazia anche se tale denominazione comprende anche figure di magistrati. Quale deve essere il compito della burocrazia ministeriale e quello della politica? Credo che il compito della burocrazia debba essere valutare tecnicamente la sostenibilità di un provvedimento, soprattutto quando si parla di provvedimenti che non sono di competenza di un certo Ministro, ma sul quale quel Ministro deve esprimere un parere.

Il burocrate può spingersi fino a dire tecnicamente che una norma è sostenibile, mai discutibile dal punto di vista politico, rimettendo alla politica l'onere di decidere. Poiché mi piace fare esempi concreti,

che per questo periodo, dall'inizio della pandemia, le aziende che hanno un debito con l'erario non soltanto si vedono sospesa la procedura di recupero, ma addirittura, contravvenendo a questa norma e in virtù dell'articolo 153 del decreto-legge 2020, hanno diritto di poter incassare i loro crediti. Non soltanto viene sospesa la procedura di recupero, ma con l'articolo 153 del citato decreto-legge possono percepire i crediti, mentre la normativa ordinaria prevede che la pubblica amministrazione prima di erogare debba accertarsi se l'azienda sia debitrice. se così è, non si capisce per quale motivo è stato respinto un emendamento che prevedeva in buona sostanza che lo stesso che lo stesso favore, in virtù di una situazione epidemiologica che ha creato tanti problemi, potesse essere applicato a quelle imprese che hanno partecipato a gare d'appalto avendo un debito magari anche inconsapevolmente con l'erario, ma che lo abbiano pagato prima dell'aggiudicazione. Non vedo qual è il problema per accettare questo emendamento che è stato segnalato dal mio Gruppo, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, ha ottenuto il parere favorevole del Ministero dell'economia e del Ministero delle attività produttive,

si è convinta che vi fosse qualcosa che non funzionava. Il primo parere di questo Ministero era che fosse apprezzabile lo sforzo, il tentativo di questo emendamento, ma esprimeva parere sfavorevole perché si viola la *par condicio.* Chiaramente abbiamo prodotto, sempre grazie alla disponibilità della vice Ministro, la documentazione che dimostrava esattamente il contrario, chiedendo una rivisitazione di quel parere. Ebbene, il secondo parere è stato peggiore del primo, quindi c'è stata una difesa sperticata di una norma che non competeva all'ufficio di diretta collaborazione del Ministro, perché cambiare le norme o decidere se le norme vanno benne o vanno modificate è compito del legislatore e non del burocrate che collabora con questo o con quel Ministro. Credo che ci sia la necessità di ritornare al primato della politica, lo dico nell'interesse del Parlamento e lo dico anche nell'interesse dell'Esecutivo. L'Esecutivo e il Parlamento non possono essere portati a passeggio dai burocrati ministeriali, ma si devono assumere la responsabilità di decidere e i burocrati si devono fermare un momento prima di quello decisionale. Personalmente, credo

sempre cortese e sempre cordiale. Lui ha detto: io sono il Ministro per i rapporti con il Parlamento e non posso non sostenere il parere di un altro Ministero, anche se non voglio entrare nel merito.

al sostegno delle imprese e delle famiglie italiane e merita sicuramente l'attenzione di questo Parlamento, del Governo e di tutti coloro che avranno a che fare con le misure attuative.

possano rinunciare all'utilizzo diretto e optare per la cessione anche parziale ad altri soggetti, tra cui istituti di credito e intermediari finanziari, anche con facoltà di successive cessioni.

Un altro aspetto positivo in tema di agricoltura è rappresentato dall'emendamento relativo all'accesso delle imprese agricole al conto termico (tema non banale, ma molto importante), che permette utilizzo degli incentivi erogati dal GSE per interventi riguardanti l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Sono state estese le produzioni della *vertical farming* e previste disposizioni in materia di prodotti di quarta gamma. Il provvedimento è importante perché va nella direzione dello sviluppo di un nuovo comparto molto innovativo e che oggi sta crescendo molto. È stata inoltre approvata la possibilità di commercializzare, fino a esaurimento scorte, i prodotti immessi in commercio o etichettati fino al 1° gennaio 2022, seppur privi dei requisiti disposti in materia di etichettatura. Ciò supera in parte le volontà precedenti. Occorrerà comunque intervenire nuovamente per risolvere le numerose questioni aperte relative agli imballaggi di numerosi prodotti (dal vino, all'olio, alle conserve). L'approvazione dell'emendamento rappresenta un elemento positivo in questo periodo di grande difficoltà per le aziende. C'è soddisfazione in tutto il settore anche per l'emendamento che prevede che per accedere agli esoneri contributivi, *ex* articolo 222 del cosiddetto i beneficiari della domanda dichiarino di non aver superato i limiti individuali fissati dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. di Stato. Anche questo è un provvedimento importante, perché va incontro all'esigenza di semplificazione espressa a gran voce dalle imprese agricole. Molti altri emendamenti hanno avuto riscontro positivo. Oltre alle luci che accenderà questo provvedimento sugli italiani, rimangono ancora delle ombre, signor Presidente, che dovranno essere assolutamente chiarite nel prossimo provvedimento. ombre che in parte oscurano oggi i volti di centinaia di migliaia di lavoratori agricoli, che con i nostri emendamenti avremmo potuto tutelare, illuminando naturalmente i loro volti da subito.

e quelli che hanno un reddito vicino alla soglia di povertà. *(Applausi)*. Noi abbiamo proposto un emendamento importante: l'indennità per i lavoratori stagionali agricoli, che mirava ad eliminare una disparità di trattamento a carico degli stessi lavoratori stagionali, sia dell'agricoltura, sia della pesca. Questi sono stati infatti esclusi dall'erogazione dell'indennità, prevista all'articolo 10 del decreto-legge per tutte le altre categorie, a cui è stata quindi riconfermata, come ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo e ai lavoratori occasionali. Volevamo con un emendamento sanare questa disparità. Non ci siamo riusciti, ma speriamo di farlo a breve. Vi è poi il sostegno ai lavoratori del comparto della trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici: proposta era finalizzata a colmare un vuoto importante, perché alla fine, con l'utilizzo della nuova assicurazione per l'impiego, non

con un sistema di investimenti che possa essere supportato dal Governo tramite Ismea. Signor Presidente, da quest'Aula oggi deve partire un messaggio chiaro al Governo e a tutto il Paese, un messaggio di ritorno alla vita. Dobbiamo riaprire, eliminare il coprifuoco e dare a centinaia di migliaia di imprese la possibilità di lavorare, di faticare, ma anche di arrivare la sera ad essere soddisfatti ed orgogliosi della propria attività. Il piano vaccinale sembra funzionare; proseguiamo su questa strada. Prima gli italiani sempre. *(Applausi)*.

ma come l'ennesima, valida spinta per la sopravvivenza dell'intero tessuto produttivo e lavorativo italiano. Come ho già sottolineato nei miei precedenti interventi in quest'Aula, il provvedimento odierno è la naturale prosecuzione del buon lavoro iniziato con il Governo Conte II. Inizialmente ci fu un decreto liquidità per dare sostegno a tutte le imprese italiane; poco prima ci fu il cosiddetto decreto cura Italia e subito dopo il decreto rilancio per supportare tutti i lavoratori italiani bloccati dalla crisi pandemica con ristori a fondo perduto. Dopo l'estate dello scorso anno arrivò il decreto agosto, seguito da quattro decreti ristori, poi confluiti in un unico testo. Non lasciammo soli i nostri cittadini e non li lasceremo soli mai, a maggior ragione adesso. Le istanze che ci arrivano quotidianamente sono due: riaperture e sostegno. Le prime stanno arrivando, seppure con la necessaria prudenza, perché nessuno ha interesse a rendere più complicata l'esistenza di chi è in difficoltà e certe strumentalizzazioni per intestarsi cose già stabilite da tutti mi indignano. Sugli aiuti si continua a lavorare giorno dopo giorno per garantire a tutti un adeguato sostegno. Come vedete, questo decreto-legge - cui seguirà anche un secondo testo di supporto economico - è una norma necessaria per la stessa sopravvivenza del nostro tessuto economico. La storia è l'unico metro di paragone a cui possiamo riferirci per valutare le azioni che stiamo compiendo. Stiamo attraversando la più grave crisi economica dal dopoguerra. Allora furono gli aiuti statunitensi con il Piano Marshall a permettere la ripartenza roboante della nostra economia; la differenza rispetto ad allora è che gli anticorpi per contrastare una crisi economica ce li siamo costruiti in casa. La costituzione di un'Unione europea forte e unita ha permesso di strutturare meccanismi che ci permetteranno di uscire da questa crisi con le nostre sole forze. Se uniamo gli sforzi economici fatti negli scorsi mesi con diversi scostamenti di bilancio ai fondi ingenti che arriveranno dall'Europa con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ecco che possiamo guardare con maggiore fiducia agli anni a venire. Anzi, voglio essere ancora più netto: dobbiamo guardare con fiducia ai prossimi mesi. Ci sono interi settori produttivi che chiedono certezze. spesso mi sono speso per portare in Parlamento le istanze del settore fieristico, e anche oggi desidero farlo lanciando, però, un monito: sappiate che se perderemo tempo, rimanendo nell'indecisione, perderemo quote di mercato a favore di piazze estere che si stanno già riorganizzando. Già abbiamo perso tempo per un'assurda crisi di Governo che grida ancora vendetta; non aggiungiamo danno a danno. Sono felice che in autunno ripartiranno grandi appuntamenti fieristici internazionali che da sempre si svolgono in Italia. A settembre riapriranno i battenti il salone del mobile di Milano e il Cersaie a Bologna: un appuntamento, quello del settore della ceramica, che conosco molto da vicino e che da sempre è stato nodale per l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Il settore ceramico vive un momento molto delicato, con i costi produttivi che salgono anno dopo anno per l'incremento del costo delle materie prime e dei pallet, che rischiano di minare la ripresa. Non ha aiutato il blocco totale per oltre un anno delle fiere nostrane e internazionali. Per settori come la ceramica e l'*export* vale l'80 per cento del fatturato. Solo dando certezze sul futuro potremo difendere questa nostra *leadership* a livello globale. Personalmente ho presentato diversi emendamenti a questo testo per sostenere il settore; sono soddisfatto che ne sia passato almeno uno, presentato anche dal collega Collina, insieme ai colleghi Croatti, Castaldi, Trentacoste, Briziarelli, Modena, Angrisani, Marinello, Parrini, Augussori, Lonardo, e supportato anche dal collega Cassese della Camera, per sostenere una nicchia, piccola ma importante: quella della ceramica artistica. L'emendamento incrementa di 2 milioni di euro il fondo previsto dal decreto-legge rilancio per sostenere il comparto della ceramica artistica tradizionale rendendo disponibili 4 milioni di euro che potranno essere utilizzati dal settore nel 2021. In un Paese come il nostro, con una tradizione artigiana fortemente radicata nei territori e una vocazione artistica importante, questa è veramente una buona notizia. Per il comparto fieristico avevo presentato anche altre due proposte che rispondevano a due diverse esigenze: due temi sui quali voglio sollecitare risposte urgenti dal Ministero dello sviluppo economico. Il primo riguarda i lavoratori dell'indotto fieristico, che da mesi sono senza stipendio e senza lavoro. Ricordo che allestitori, comparto sicurezza, falegnameria - solo per citarne alcuni - impiegano personale con contratti di varia tipologia spesso a chiamata diretta solo per gli eventi. La seconda necessità da valorizzare è l'attrazione dei visitatori esteri interessati a partecipare ad eventi fieristici sul nostro territorio. Come già sottolineato, è dall'estero che questo settore trova gran parte del proprio sostentamento. Come MoVimento 5 Stelle abbiamo sempre sostenuto l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Il ministro Di Maio ho sempre investito su questo; spero che il Governo voglia continuare su questo sentiero. Cito anche un'altra proposta emendativa approvata a questo testo, una norma per valorizzare l'ambiente e ridurre speculazioni economiche su di esso. un emendamento che esclude dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica, alimentati a biogas e biomasse, nonché gli impianti per la produzione di biometano che siano in infrazione rispetto alle normative europee o che facciano approvvigionamento di materie prime in territori diversi dal Paese. Colleghi, concludo auspicando che in Assemblea ci sia la più ampia convergenza sull'approvazione del testo abbiamo licenziato l'ennesimo scostamento di bilancio: nessuno può sottrarsi dal trasformare quello scostamento in aiuti rapidi e concreti. Il nostro unico obiettivo deve essere quello di dare risposte concrete agli italiani, ai lavoratori e alle imprese. Dobbiamo rendere più solide le fondamenta del nostro sistema produttivo. Oggi siamo chiamati a governare e a superare questa crisi, con una visione a lungo termine: perdere tempo sarebbe imperdonabile.

Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, a vedere la somma totale degli scostamenti fatti, tremano veramente i polsi, perché 156

ci siamo sempre preoccupati parecchio, più che dello scostamento, di dove queste risorse sarebbero state allocate. Come tutti ricorderanno, non abbiamo espresso sempre un parere così entusiasta nei confronti del lavoro del precedente neppure di quello di prima ancora, eppure non eravamo in pandemia. Confermiamo questa preoccupazione, perché

Non l'abbiamo apprezzato perché, se andiamo a vedere esclusivamente quanto è arrivato nelle tasche degli imprenditori in tutto questo anno difficile, alle nostre spalle - parlerò poi più approfonditamente di quello che abbiamo di fronte, per quanto riguarda il futuro

tutte le aziende, non certo quelle decotte, come ogni tanto ci ricorda il presidente Draghi, ma quelle che hanno avuto, nel recente passato, i problemi di tutte le imprese italiane, le difficoltà con l'erario, talvolta l'impossibilità di pagare tutto quello che c'era da pagare, perché a un certo punto si sono trovate nella necessità di scegliere tra pagare gli stipendi ai propri dipendenti o pagare le tasse.

ha perso la voce a forza di sostenere il mondo produttivo. Quando per due anni e mezzo abbiamo parlato di sviluppo, di impresa e di lavoro, venivamo guardati come extraterrestri.

come del resto i nostri componenti della Commissione bilancio, uno per tutti il capogruppo Damiani. Ogni volta ci troviamo in Commissione a spiegare quanto è importante sostenere uno dei settori fondamentali dell'economia nazionale come il turismo, per esempio. Ci siamo dovuti ammazzare per fare una battaglia, per esempio, sui bus turistici per 20 milioni di euro, quando abbiamo buttato centinaia di milioni di milioni da altre parti, dove forse servivano meno che in questo caso. Abbiamo dovuto spiegare per settimane che aziende come quelle del turismo non lavorano da Abbiamo dovuto spiegare che i bus sono fermi nei piazzali e costano. Abbiamo dovuto spiegare che i servizi scolastici aggiuntivi per i trasporti sono stati insufficienti in termini numerici ed economici e, quindi, dovevano essere sostenuti. Abbiamo dovuto lottare per spiegare quanto le strutture ricettive che erano chiuse avrebbero dovuto avere agevolazioni. Siamo arrivati a dei risultati: siamo arrivati

Lo Stato e i funzionari facciano il loro mestiere; alla politica ci pensiamo noi, che rispondiamo direttamente agli italiani, i quali non fanno sconti e fanno bene. Quando protestano, hanno tutto il diritto di farlo. È possibile che un senatore della Repubblica si debba mettere a litigare con un funzionario dello Stato su una posizione politica e non tecnica? Non ha senso; non va bene e non si deve fare così.

Il lavoro è sufficiente e ha una prospettiva positiva. Il prossimo decreto sicuramente sanerà queste lacune, ma non ci dimentichiamo il ruolo centrale che deve avere la politica rispetto al sistema della burocrazia. Noi abbiamo il diritto di decidere, gli altri hanno il dovere di eseguire. Se perdiamo di vista questo passaggio, allora vuol dire che è inutile rimanere qui in quest'Aula. Signor Presidente, abbiamo sentito dai relatori tutto quanto di buono è stato fatto in questi giorni, in Parlamento e dal Parlamento. Ecco, questa è già una differenza rispetto a quanto accadeva con il precedente Governo. Vede, signor Presidente, il presidente Draghi ci ha richiamato al fatto che il Governo è il Governo degli italiani. Bene, noi abbiamo dimostrato in questi giorni che anche il Parlamento è il Parlamento degli italiani.

della somma dei primi 32 miliardi cui assommano le misure contenute dal primo dei decreti sostegni. Dico i primi 32 miliardi perché ce ne saranno altri 40. La somma complessiva è di 72 miliardi, pensati in una logica complessiva, pensati in maniera organica. Questo è un passaggio fondamentale. Era quello che, come Lega, ci eravamo impegnati a fare anche nei provvedimenti ed è quello che stiamo facendo. Già il passaggio del nome, da decreto ristori a decreto sostegni, la dice lunga su quale sia il passaggio di impostazione, che il Paese ci chiedeva e che noi stiamo attuando. Matteo Salvini ha annunciato il sostegno al Governo, lo ha fatto con due punti fermi e chiari: il cambio di prospettiva e il cambio di passo.

un cambio di passo e di prospettiva c'è stato sulle riaperture, che sono finalmente iniziate, con quel rischio calcolato, che non è incoscienza e che ha un'incidenza diretta anche sulla portata economica dei provvedimenti. tanto più le aziende potranno tornare a lavorare (il sostegno migliore che si può loro dare), tanto più si potranno concentrare le risorse su chi ancora dovrà soffrire prima di poter riaprire. Sui *social* è comparso da qualche ora un *post* in cui ci si lamenta e ci si preoccupa del fatto che questa mattina sia stata bocciata l'estensione del coprifuoco a marzo, al passato. Noi, invece, ci preoccupiamo di aver ottenuto, come Lega, il fatto che a maggio, fra pochi giorni, si potrà rivedere l'orario delle aperture, se i dati lo consentiranno. *(Applausi)*. Dati che, è bene ricordarlo, devono essere richiamati in negativo, purtroppo, quando serve, ma devono valere, perché la scienza vale sempre e non a corrente alternata, quando si potrà dire, come si può dire in questi giorni, che i dati migliorano e che questo permetterà le riaperture. vale per l'entità delle risorse. Facevo prima accenno ai 40 miliardi già stanziati e già impegnati, in parte, per il prossimo decreto e, ovviamente, sull'utilizzo delle risorse. In questo decreto sostegni non troverete neanche un euro speso inutilmente per monopattini o quant'altro. Noi, responsabilmente, tutti insieme, abbiamo impiegato fino all'ultimo centesimo pensando al debito che stiamo contraendo con i nostri figli. Qui c'è il cambio di passo

che ci animerà anche nei prossimi mesi. Purtroppo, non abbiamo la versione in francese e neanche in tedesco. L'abbiamo solo in italiano, perché è pensato per gli italiani. È un metodo che punta a sostenere il Governo, ma a farlo in maniera leale e propositiva. Qualcuno, pensando di offenderci, ha descritto la Lega come un partito di lotta e di governo. Ebbene, non è un ossimoro, ma una naturale conseguenza. Noi siamo orgogliosi di essere un partito di lotta e di governo perché i cittadini, le famiglie e le imprese stanno lottando per arrivare alla fine del mese, per uscire da questa crisi ed è doveroso che i rappresentanti dei cittadini lottino per trovare delle soluzioni, si impegnino per convincere i compagni di viaggio che abbiamo in questo sostegno al Governo della necessità di fare sempre qualcosa di più nell'interesse dei cittadini. Il testo base del decreto-legge aveva già superato problemi enormi. Si tende a dimenticare (ce lo siamo scordati) il sistema dei codici Ateco, che tanto vigliacco e ingiusto era stato per molte imprese. grazie a questa maggioranza e all'impegno della Lega che già nel testo base quel sistema dei codici Ateco, che era il cardine negativo del decreto ristori, è stato sistemato. abbiamo lavorato per l'esenzione dal pagamento del canone RAI, per i contributi alle associazioni, per il riconoscimento della lingua dei segni (eravamo l'ultimo Paese in Europa a non aver fatto nulla per questo); abbiamo lavorato per i lavoratori fragili, per completare quel periodo di cassa integrazione non coperto. Sono tutte misure proposte dalla Lega, ma condivise da tutti e questa è un'altra grande differenza. modo sono state condivise da tutti le misure a sostegno del comparto della ceramica (il collega Lanzi ha ricordato tutti i senatori che hanno sottoscritto quel provvedimento, tra i quali c'erano ovviamente anche i senatori della Lega); così come sono state condivise le misure a sostegno delle città città d'arte minori e dei borghi minori per dimensione (10 milioni di euro). Sono tutte misure condivise, non una somma di singoli interessi portati dal singolo partito, ma un unico interesse generale. Questa è la grande differenza che richiamava anche il collega Manca in apertura:

fra pochi giorni con gli ulteriori 40 miliardi, perché diventino risposte da qui a poco. Non abbiamo voluto il solito ordine del giorno e non a caso, lavorandoci insieme notte tempo, abbiamo individuato 11 punti che vorrei ricordare rapidamente e che

come è giusto che un Parlamento faccia, a impiegare le risorse dello scostamento per ulteriori contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA e di tutte le imprese dei diversi settori sulle quali si è abbattuta la crisi Covid; a individuare adeguate misure di sostegno per le imprese ad alta intensità di lavoro (le mense, i servizi di pulizie, eccetera), con particolare riguardo alle misure per la cassa integrazione; a individuare misure finalizzate a sostenere l'erogazione del credito delle piccole e medie imprese (PMI) e a prorogare fino al 31 dicembre 2021 la

allo stanziamento di adeguate risorse, pari almeno a 600 milioni di euro, in favore degli enti locali, da destinare alla riduzione del pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) da parte delle imprese; allo stanziamento di ulteriori risorse, pari almeno a 100 milioni di euro, in favore del fondo per la montagna, di cui all'articolo 2 del decreto-legge attualmente in esame; alla proroga delle indennità a favore di lavoratori stagionali, con particolare riguardo ai lavoratori stagionali in agricoltura, del settore del turismo, dei lavoratori ciclici dello spettacolo e della cultura; allo stanziamento di risorse aggiuntive in favore degli enti locali; allo stanziamento di adeguate risorse per affrontare il disagio psicologico dei minori. Abbiamo impegnato il Governo per misure finalizzate a risolvere il problema del settore fiere, come già altri hanno ricordato, e per misure in favore delle imprese che gestiscono attività di servizi culturali, eventi, congressi, spettacoli, cinema, teatro, al settore del *wedding.* Ebbene, non è un elenco, ma è quello che noi chiediamo ai cittadini di andare a spuntare sul prossimo decreto-legge per dimostrare che questa classe politica ha dignità e rispetto del Paese. Quelle cifre le troveranno, perché questo impegno noi lo manterremo da qui ai prossimi mesi. *(Applausi)*.

un ascolto delle categorie audite e delle loro puntuali istanze portate nelle Commissioni riunite 5a e 6a del Senato, che ha visto l'accoglimento di molte proposte; ma soprattutto un confronto pieno tra tutti i Gruppi parlamentari in Commissione e un ascolto attento da parte dei relatori Manca e Toffanin. E siccome sono di parte, ci tengo in particolare a ringraziare la senatrice Toffanin, che ha sposato in pieno il ruolo di relatrice seguendo con passione e competenza, punto per punto, l'evolversi del testo nelle Commissioni riunite. Il decreto-legge e le disposizioni attuative che lo accompagneranno hanno l'importante compito di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del Covid-19 e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. utilizza per questo scopo 31 miliardi rimasti nel primo scostamento deliberato dal Parlamento e traccia anche la strada per il prossimo decreto-legge sostegni-*bis*, che dovrebbe vedere la luce la prossima settimana e che metterà in campo gli altri 40 miliardi dell'ultimo scostamento, o comunque buona parte di essi, da destinarsi, come avete detto precedentemente, a quei ristori per altrettante categorie che oggi non hanno potuto avere una loro soddisfazione. Su questo ritengo ci sia l'impegno del Governo affinché si colmi tale lacuna. dicevo, alle imprese arriva un bel po' di ossigeno: 11 miliardi di contributi a fondo perduto e circa 15 miliardi di aiuti. Al lavoro e al contrasto alla povertà vanno 6 miliardi; alla salute e alla sicurezza circa 3 miliardi e mezzo, investendo sui vaccini con una campagna che procede spedita grazie al generale Figliuolo, all'organizzazione messa in piedi, ed inoltre alle risorse di farmaci anti-Covid. Soprattutto, quello che ci piace è l'organizzazione nuova del generale Figliuolo, che sta avendo dei successi importanti: oltre 500.000 vaccinati ogni giorno sono la vera speranza di poter allontanare lo spettro di questa pandemia. Agli enti territoriali sono andati 3 miliardi e mezzo, con i quali potranno anche potenziare il trasporto pubblico locale, che è il vero punto debole della lotta alla diffusione del virus. È stato dato largo spazio, come dicevo, anche alle modifiche parlamentari: innanzitutto tengo a citare l'esenzione della prima rata IMU da me sostenuta insieme ai colleghi di Forza Italia), ed altri emendamenti aggiunti che hanno una copertura di 216 milioni di euro. Si tratta di un sostegno per andare incontro a quei soggetti che, già colpiti dalle chiusure e quindi da mancati ricavi, verrebbero pure penalizzati da una tassa per dei beni immobili che nel periodo non hanno prodotto un reddito, in quanto le attività che vi si svolgono erano ferme. Per parte mia, ho anche soddisfazione per una misura a cui tenevo molto: l'incentivazione del *welfare* aziendale. Ci credo e spero che sarà presente anche nel prossimo decreto-legge sostegni con una cifra superiore a quella destinata da questo provvedimento. stesso modo, sono soddisfatto dell'approvazione della norma che riguarda il Porto canale di Cagliari, dove è già in corso un processo importante di riconversione industriale, che va accompagnato, in particolare adesso, proprio per tutelare le diverse centinaia di posti di lavoro interessati dalle crisi aziendali e restituire centralità al porto industriale di Cagliari. Naturalmente, su questo tema, non c'è solo

e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, deliberata più di un anno e mezzo fa dal Senato. Lo dobbiamo

Signora Presidente, signora Sottosegretario, questo è un provvedimento davvero decisivo e importante, di cui il relatore Manca ha sottolineato alcuni aspetti che noi condividiamo in maniera particolare. Siamo entrati nella fase dei sostegni; non è solo un fatto nominale, ma significa che l'economia del Paese si avvia verso una ripartenza

quali attività e di quali lavori si svolgono o non si svolgono in questa Aula. L'impegno principale di queste settimane in Senato - forse è bene ricordarlo a tutti - è stato un enorme impegno economico,

però noi affrontiamo quella parte fondamentale per la ripresa di questo Paese che riguarda la scuola, la cultura, il settore della ricerca e dell'università e, in ultima analisi, anche lo sport, un tema di cui tante volte io colpevolmente mi occupo un po' meno, tra le tante materie della nostra Commissione. Quest'Aula e questa maggioranza così composita

vengono stanziati, con il voto che esprimeremo nelle prossime ore, per le società sportive dilettantistiche. Si tratta di un impegno importante e di una scelta rilevante del Parlamento in termini percentuali di spesa. Ovviamente è una quantità contenuta rispetto ai bisogni effettivi di questo mondo, che è stato colpito pesantemente dalla pandemia, perché ha avuto il blocco delle attività e anche un aumento significativo delle spese, dovendosi riorganizzare completamente e dovendo

ma come lo sport diffuso per tutti che diventa una pratica quotidiana. Si tratta di una scelta molto importante. Ci sono altri interventi che sono stati approvati dei tanti che avevamo provato a proporre. Ad esempio ve n'è uno molto importante di

di riconoscere quella funzione e di riconoscere un credito, sostenendo una ripresa. In questo senso va anche un altro emendamento che proroga la funzione dei *voucher*;

concretizzare il loro acquisto, vanificato dal Covid, in un tempo in cui lo potranno fare in tranquillità e in serenità e la proroga fino a trentasei mesi dà questo spazio, ma onestamente questo vuol dire anche permettere a tutto quel mondo di riorganizzarsi

nei confronti dei Comuni, facendo in modo che non sia a spese loro. Per concludere il punto è che noi siamo seriamente impegnati a tendere una mano, tentare di coprire

Presidente, desidero innanzitutto ringraziare moltissimo i relatori, in primo luogo la relatrice Toffanin per il lavoro che ha svolto, il relatore Manca, i colleghi della Commissione, a cominciare dal Capogruppo, perché effettivamente si è cercato di fare un lavoro positivo, tenendo come sempre conto delle condizioni date. Credo che possiamo partire proprio da queste condizioni date per fare una breve analisi.

un decreto-legge che parzialmente riusciva a dare delle risposte ed è vero, nel senso che sicuramente un quadro più completo lo si avrà con l'approvazione del cosiddetto decreto sostegni-*bis*. Va anche detto che sono state introdotte alcune modifiche importanti, quelle ad esempio relative al fatturato o anche relative al mezzo di pagamento, perché non so se avete notato che non si parla più

da quelle parole che inizialmente disse il presidente Draghi qui, parlando del coinvolgimento dell'Esercito e della Protezione civile, che sarebbe riuscito nel giro di due mesi e mezzo a portarci al livello a cui ci ha portati in termini di campagna vaccinale. Non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché questo è il primo motivo per cui siamo - pur diversi - insieme, perché stiamo salvando,

le questioni che si è riusciti ad affrontare. Altre sono rimaste indietro, ne siamo rammaricati e consapevoli, ma

ad esempio in materia di disabilità, contribuendo alla Federazione nazionale delle istituzioni *pro* ciechi, abbiamo dato risposte alle esigenze dei Comuni con la fondazione ANCI per gli impianti sportivi, cosa che aiuta i Comuni, soprattutto i più piccoli. Abbiamo cercato di dare delle risposte al problema delle città santuario. Come sapete, in

altrimenti avremmo dovuto avere un *plafond* e una capacità di manovra sicuramente maggiori. È poi chiaro che tutte le forze politiche, nel momento in cui fanno

finalmente ha cominciato a sentir parlare di impresa in un certo modo. Ciò è vero e sicuramente da questo punto di vista siamo riusciti a dare un apporto positivo: imprese, libere professioni e altro ancora.

le condizioni di lavoro migliori che potevamo dare al Paese, anche in termini di linee e indirizzi da perseguire.

Governo, onorevoli colleghi, ho gestito la mia prima attività di partita IVA a diciassette anni. Formalmente risultavo dipendente, ma sostanzialmente gestivo io l'attività, fino a che non mi sono diplomato e ho potuto intestarmi la licenza senza dover sostenere l'esame alla Camera di commercio (cosa che all'epoca era possibile).

garantiti, di partite IVA e di coloro che sono sempre stati gli ultimi nell'attenzione dei Governi precedenti so perfettamente di cosa sto parlando. Ho contezza di cosa significhi

e purtroppo, come tutti sappiamo bene, hanno avuto come conseguenza diretta dei morti e delle vittime, a cui inevitabilmente va il primo pensiero.

qualcuno ha smesso di lottare e deciso di porre fine alle proprie sofferenze rinunciando addirittura alla propria vita. Questo lo dico perché voglio evidenziare che una delle conseguenze

che, provati dalla difficoltà di affrontare una situazione così complessa e pesante, non riescono ad andare avanti. Questo succede dopo un terremoto, dopo dopo una pandemia e succede perché spesso non si tiene conto di un elemento che, a differenza di tutti gli altri, è parzialmente nel controllo di tutti noi; mi riferisco al tempo, che se perso e se non investito proficuamente, se non finalizzato ad uscire dalla difficoltà nel minor arco temporale possibile, rischia di diventare quel rimpianto per cui si arriva a fare la cosa giusta, ma non ha l'effetto desiderato, perché la si è fatta troppo tardi. Quindi, colleghi, la prima domanda che mi viene ora è: vogliamo veramente arrivare a rimpiangere il fatto di non essere arrivati in tempo? *(Applausi)*. Ricordo una barzelletta di tanto tempo fa che diceva: «L'operazione è riuscita perfettamente, ma il paziente è morto». *(Applausi)*. Noi non vogliamo che il paziente noi vogliamo che le misure messe in campo, che spesso sono utili, opportune ed efficaci, non siano vanificate dal fattore tempo, che è l'unico che in parte possiamo controllare. Ecco perché la Lega si sta impegnando, per anticipare le riaperture; non perché vogliamo contrapporci all'azione del Governo, ma perché da pragmatici e da persone responsabili abbiamo fatto la valutazione di tutte le alternative. Quindi, riflettendo per alternative e non in termini assoluti

ad applicare quelle misure di buon senso che chiediamo, sarebbero di gran lunga inferiori al rischio di non farlo. Noi non vogliamo mitigare le misure di cautela, ma vogliamo evitare che la cautela diventi eccessiva e che le conseguenze della stessa portino a problemi ulteriori. Come dicevo prima, in questo decreto-legge ci sono passi nella giusta direzione. Questo non significa che il percorso si è concluso (lo sappiamo bene noi e lo sa altrettanto bene il Governo, che infatti sta già lavorando al decreto successivo), ma questi passi innegabilmente ci sono. Da marchigiano non posso che essere soddisfatto delle misure a favore delle Regioni colpite da emergenze. Da terremotato non posso che essere soddisfatto per le misure previste per le nostre zone. Da ex sindaco non posso che esprimere soddisfazione per le misure previste a favore dei Comuni e da montanaro esprimo la mia piena soddisfazione per quanto previsto per le attività Vengo da un comprensorio sciistico, che è stato colpito duramente prima dal terremoto e poi dal Covid, ma mi ha insegnato quanto sia importante il turismo invernale quanto siano importanti le stazioni di risalita, non solo per il fatturato diretto che generano, ma anche per tutto l'indotto che per le zone di montagna spesso è vitale. Oltre alle misure che ho poc'anzi indicato, la mia soddisfazione va anche come ho evidenziato prima - per le partite IVA, categoria a cui mi sono pregiato di appartenere per la stragrande maggioranza della mia vita. Mi riferisco all'esenzione della prima rata IMU, al contributo diretto ai liberi professionisti, sempre e sistematicamente ignorati da tutti, che invece abbiamo riportato prepotentemente all'attenzione di questo Parlamento e del Governo; quei liberi professionisti che costituiscono l'ossatura economica del nostro Paese, che pagano le tasse, che generano milioni di posti di lavoro che non venivano mai considerati. Concludo come avevo iniziato: finalmente gli ignorati, finalmente i dimenticati, finalmente coloro che non avevano mai avuto l'attenzione da parte del Governo sono ritornati prepotentemente sotto ai riflettori come meritavano,

È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà. Non posso che giudicare insufficienti le risposte che sono state date da questo decreto-legge sostegni, che fanno il paio sia con le misure restrittive sia con le claudicanti riaperture che hanno messo e mettono a rischio la sopravvivenza anche di tante imprese. Non è razionale sostenere che si può salvare un'impresa dandole

Uno degli strumenti importanti, forse l'unico che aveva portato avanti bene questo Governo, era legato al superbonus del 110 per cento. È sicuramente uno strumento importante che serve per aiutare e può essere un volano per la nostra economia nazionale, oltre a rappresentare uno strumento strategico per raggiungere gli obiettivi della rigenerazione urbana. È quindi uno strumento che non deve essere assolutamente perduto, ma è un'occasione che va colta. Come dicevo poc'anzi, deve essere un volano per l'economia nazionale, tanto è vero che abbiamo visto negli ultimi mesi come questo strumento abbia

e, solo dopo dieci giorni, siamo arrivati a un incremento di quasi il 40 per cento, passando a 9.207 interventi, per un valore di oltre un miliardo. il superbonus rappresenterebbe una misura anticiclica. Fratelli d'Italia ha sempre ritenuto che, per rilanciare l'economia, e soprattutto per sostenere le imprese, fosse necessario incentivare i consumi e anche la produzione. Questa è la logica che di fatto sottende anche al superbonus; ma per poter arrivare a questo sono fondamentali due elementi: il primo è la proroga. È fondamentale una proroga al 2023

Anche in questo caso il Governo ha annunciato, qualche settimana fa, il decreto-legge semplificazioni; quindi, sarebbe importante che il superbonus rientrasse in questa logica di semplificazione. Soltanto da un punto di vista verbale c'è stato un impegno da parte del *premier* Draghi sia per quanto riguarda la proroga sia per quanto concerne il discorso della

nel campo dell'edilizia, che rappresentano un asse portante della nostra economia. Quindi vigileremo, affinché queste parole si possano realizzare in atti concreti.

Manca e Toffanin e dal Governo, perché il decreto-legge sostegni, che ha rappresentato l'esordio del Governo Draghi in materia di misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, è potuto essere migliorato dalla fase emendativa, sviluppata dalle Commissioni. Ovviamente non bisogna dimenticare la base di partenza, ovvero il testo del decreto-legge tuttora in vigore, che contiene misure finanziate dall'ultimo scostamento di bilancio presentato dal Governo precedente, di 50 miliardi di euro in termini di cassa, che il Governo Draghi, nella sua composizione largamente rappresentativa delle forze politiche parlamentari, ha interpretato in modo adeguato.

non ci ha aiutato a fare delle valutazioni complessive, che preventivamente potessero consentirci di dare delle risposte mirate. Oggi però, dopo un anno, le valutazioni sulle priorità per salvaguardare il sistema produttivo ed aiutarlo a mettersi non solo in sicurezza, ma anche nelle condizioni di ripartire, sono più precise. Ci siamo infatti concentrati sul sollevare le imprese, in modo particolare i pubblici esercizi, da quei costi fissi che in questo momento dell'anno avrebbero rappresentato un problema difficilmente sopportabile. Penso all'esenzione della prima rata dell'IMU, all'esenzione del canone unico per ambulanti al canone RAI per i pubblici esercizi, all'eliminazione dell'Irpef per i canoni sugli affitti non percepiti, alla proroga a settembre del versamento IRAP. Questi sono i principali interventi che il lavoro parlamentare ha potuto aggiungere al testo del decreto-legge, ma chiaramente ciò non può essere sufficiente. Le esigenze sono evidenti e, insieme anche agli altri Gruppi parlamentari che le hanno condivise, le abbiamo riassunte in un ordine del giorno impegnativo per il Governo e ci attendiamo di vederle già inserite nel prossimo imminente decreto-legge, che è chiamato a mettere a terra l'ulteriore dotazione di 40 miliardi di euro, relativi allo scostamento di bilancio votato dieci giorni fa. rappresentano i contenuti, che riteniamo possano completare questo lungo anno di rincorsa rispetto alla pandemia, per tamponare gli effetti negativi sul sistema economico e che voglio citare in sintesi. prorogare almeno fino alla fine del 2021 la concessione di garanzie statali sui prestiti del fondo di garanzia PMI e Sace e, in tale ambito, appare necessario l'allungamento almeno da sei a quindici anni della durata delle garanzie statali su prestiti maggiori di 30.000 euro. prorogare la moratoria su mutui e prestiti, che riguarda 173 miliardi di euro di prestiti in scadenza a fine giugno 2021, molti dei quali rischiano di diventare sofferenze bancarie, in ragione della mancata ripresa dell'attività e del lavoro; in tale ambito appare opportuno valutare anche un allungamento delle rate di restituzione di mutui e prestiti, di sei mesi se di quota capitale più interessi e di dodici mesi se limitata alla quota capitale. gli aiuti alle imprese e la nuova tornata di ristori, da affiancare a quelli del primo decreto sostegni, con l'invio automatico a chi ha ottenuto i ristori del primo decreto e con una consistente maggiorazione per le attività chiuse per legge. nuove misure per compensare i costi fissi delle imprese, sul modello già sperimentato in altri Paesi dell'Unione europea, per affitti commerciali, bollette elettriche, spese di sanificazione e Tari, insieme ad altre misure specifiche. Bisogna prevedere un intervento significativo relativamente alla decontribuzione per assunzioni stagionali in particolare nel settore turistico ricettivo; un completamento degli interventi di aiuto alle famiglie per la lotta alla povertà, con particolare riguardo al rifinanziamento della flessibilizzazione del fondo comunale di solidarietà, alimentare e sociale per tutto il 2021. Occorre incrementare le risorse destinate alla montagna; stanziare adeguate risorse finalizzate ad affrontare le problematiche del disagio psicologico dei minori conseguenti all'emergenza Covid-19; predisporre misure finalizzate a risolvere problematiche del settore fiere; prevedere misure in favore delle imprese che gestiscono attività e servizi culturali (eventi, congressi e spettacoli cinematografici, teatrali, compreso il loro indotto) oggetto di chiusura in ragione dell'emergenza sanitaria Covid-19, con particolare riguardo all'esenzione dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di apertura di suddette attività.

rappresentano un impegno cui il Governo deve assolvere. Un ultimo passaggio lo voglio dedicare al mondo della cooperazione, che attraverso le tante cooperative sociali ha rappresentato in tanti territori un pilastro del terzo settore, che si è fatto carico di attutire gli impatti economici e sociali della pandemia. La rete delle cooperative sociali rappresenta nel nostro Paese un esempio concreto non solo di solidarietà, ma anche di resilienza. Se posso dire, tutta la cooperazione nel suo complesso rappresenta nel nostro Paese un esempio concreto non solo di solidarietà, ma anche di resilienza perché anche le cooperative di produzione e lavoro, quelle di consumo e di servizio, le coop agricole e di trasformazione dei prodotti hanno saputo adattarsi, pur con tante difficoltà, a questo anno terribile. Con alcune norme aggiuntive abbiamo dato la possibilità a questa realtà di predisporsi meglio alla ripresa, che queste settimane di vaccinazione a ritmo sostenuto ci fanno vedere più vicina.

soprattutto per il mondo dello spettacolo. Prima il senatore Collina parlava del mondo del sociale. So bene ciò che fa perché vengo dal mondo del sociale. Loro hanno continuato comunque a lavorare. Credo che, invece, dobbiamo dare più attenzione e intervenire al più presto sul contrasto alla povertà in una maniera diversa. Bisognerebbe dare più sostegno agli enti territoriali perché essi, insieme ai sindaci, sono tutti in difficoltà. Se aiutiamo gli enti territoriali, automaticamente aiuteremo le attività che in questo periodo - parlo dei piccoli artigiani - sono stati in grave difficoltà. Nonostante tutto, le piccole imprese hanno continuato a pagare la Tari, come hanno continuato a pagare l'occupazione del suolo pubblico. Faccio un esempio banale, ma serio e vero. I parrucchieri hanno tenuto le loro attività chiuse, ma nonostante questo hanno continuato a pagare i rifiuti speciali. Faccio questi esempi perché, se aiutiamo tutti gli enti e le nostre città, automaticamente queste persone possono essere aiutate. Sulla campagna vaccinale, nulla da dire. Il generale Figliuolo sta portando a termine gli obiettivi che tutti quanti ci eravamo imposti. Io, però, vorrei porre l'attenzione, in particolare, sulla questione del credito di imposta di industria: questo è l'obiettivo del mio intervento. I crediti d'imposta possono essere utilizzati non necessariamente in compensazione, ma anche ceduti a soggetti terzi, tra i quali anche istituti di credito e intermediari finanziari. Questa opzione riguarderebbe solo i crediti maturati dalle imprese in relazione agli investimenti in beni strumentali, sia quelli del 4.0 sia quelli tradizionali. In questa maniera, daremmo anche nuovo ossigeno e nuovi investimenti soprattutto all'agricoltura, che non è risultato da poco. Questa è un'ottima iniziativa che - a mio parere - potrebbe essere intesa anche per quanto concerne il credito di imposta e per i *bonus* relativi agli investimenti per il Mezzogiorno. Se la *ratio* del *recovery plan* è aiutare le zone più in sofferenza, non vedo perché non estendere questa possibilità alle misure di riferimento.

e si possa dare così alle imprese la possibilità di effettuare ulteriori investimenti con più serenità, visto che in questo periodo la serenità è stata loro

Signor Presidente, colleghi, il mio intervento sarà riferito a una sola categoria tra le tante di cui si occupa questo decreto: i lavoratori fragili. fragili? Sono, prima di tutto, persone che hanno la sfortuna di avere una fragilità, sono persone deboli. Stiamo parlando di persone immunodepresse, trapiantate o con disabilità gravi che, per un anno, hanno dovuto dividersi tra la scelta del lavoro e la scelta della salute. Nei primi mesi della pandemia, fino a metà ottobre, per non esporli al contagio, coloro che non potevano essere assegnati al lavoro agile potevano essere collocati in malattia, parificata al ricovero ospedaliero, anche se con garanzie diverse da contratto a contratto. Poi, però, essi sono stati abbandonati dal Governo Conte fino al 31 dicembre, proprio durante la seconda ondata; costretti a tornare al lavoro, magari in luoghi affollati, e i più sfortunati andandoci con un mezzo pubblico. Si è detto che ciò è avvenuto per mancanza di fondi. Ma com'è possibile? Com'è possibile che un Governo non abbia trovato le risorse per salvaguardare persone così fragili e, invece, quei fondi li abbia trovati per i monopattini e per i banchi a rotelle? Ancora coperti, ma solo per i mesi di gennaio e febbraio, e poi di nuovo il vuoto, in un tira e molla continuo che, oltre ai rischi sanitari, ha esposto questi lavoratori ad uno sconforto e ad uno stato di preoccupazione continuo, altrettanto nocivi per la loro salute. Solo la Lega si è battuta, per mesi, per dare ascolto e quindi risposte a queste categorie. Da marzo, finalmente, con il nuovo Governo abbiamo agito subito e siamo riusciti ad ottenere, con questo decreto, che le tutele venissero estese fino al 30 giugno. Abbiamo sanato, in modo retroattivo, il buco normativo dal 15 ottobre al 31 dicembre. E, soprattutto, abbiamo reso vincolante per tutti il non impatto sul comporto a partire dal 17 marzo 2020, inizio della pandemia. Si conclude oggi, con successo, una battaglia che ci ha visto, spesso, unica voce nel deserto. Ho perso il conto di quanti interventi ho tenuto in quest'Aula e in Commissione e di quanti emendamenti e ordini del giorno ho presentato. Mi sono scontrato sempre contro un muro di gomma posto da chi diceva di comprendere le esigenze, ma nulla faceva. Queste persone sono le stesse che oggi si autocelebrano e cercano vergognosamente di intestarsi la norma e il buon esito della vicenda. È proprio vero che la vittoria ha tante madri, mentre la colpa è sempre orfana. Dico chiaramente che, solo grazie alla Lega e alla tenacia di due sue fantastiche donne,

Per loro fortuna ci siamo noi dalla loro parte, dalla parte dei fragili, dei deboli e degli ultimi, quelli che voi avete dimenticato.

Signor Presidente, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Questo sintetizza a pieno il pensiero che oggi gli italiani hanno dell'Esecutivo in carica. Abbiamo dovuto assistere a una crisi di Governo nel pieno dell'emergenza perché, per stessa ammissione degli alleati, il precedente Governo era ormai ad una deriva irrecuperabile. È nato il nuovo Governo Draghi e le forze politiche che lo compongono lo hanno trionfalmente autoproclamato Governo dei migliori, facendo credere agli italiani che ormai potevano stare tranquilli, perché sarebbe cambiato tutto. Purtroppo così non è stato e in solo due mesi gli italiani si sono resi conto che tutte le rassicurazioni che erano state loro propinate sul cambio di passo sono risultate vane: hanno cambiato tutto, ma nella sostanza non è cambiato ancora nulla. Ancora una volta riemerge l'antico vizio di frammentare in tanti rivoli i circa 50 miliardi necessari per la copertura finanziaria del decreto-legge che si disperdono in tanti nuovi fondi di scarso effetto moltiplicatore sulla crescita. Ormai è chiaro: ciò che conta è buttare fumo negli occhi con *bonus* e ristori, che poi ristori non sono e che certamente non possono rappresentare delle misure strutturali di cui il nostro Paese ha bisogno. Le manifestazioni di protesta di questi giorni ne sono la riprova.

che, anche a causa della cervellotica azione multicolore sulle aperture e chiusure delle Regioni, sta compromettendo la sopravvivenza di tante realtà economiche. Basti pensare a un esempio pratico: in caso di perdite di esercizio pari a 60.000 euro, nelle casse dei professionisti e partite IVA arriveranno appena 3.000 euro; senza parlare poi dei professionisti che, in base a quello che viene loro riconosciuto, prenderanno solo poco più di 1.000 euro. A preoccupare ancora di più sono le categorie sociali produttive, che sono rimaste inascoltate. I numerosi emendamenti presentati da Fratelli d'Italia non sono valsi a nulla. Come forza di opposizione intransigente, ma anche pronta a offrire il proprio contributo in termini propositivi, tese a ottenere ristori proporzionati alle perdite; la moratoria fiscale per almeno due anni; il taglio del cuneo fiscale; il pagamento di *bonus*; ristori e indennizzi sospesi; l'eliminazione del *cashback.* Tuttavia non siamo stati ascoltati. Se si continua su questa linea, il nostro Paese è destinato al *default*, perché sarà impossibile riattivare l'economia nazionale, tenuto conto che nel frattempo le piccole e medie imprese e i commercianti, senza reali sostegni di liquidità e indebitati come non mai, si ritroveranno a dover pagare i costi fissi e le utenze, che nel frattempo sono incomprensibilmente aumentati, con con evidente responsabilità del Governo, che non è intervenuto prontamente nei confronti delle grandi aziende di distribuzione. Continueremo a pagare una tassa dopo l'altra senza alcuna prospettiva di un ritorno concreto alla normalità. Senza considerare che ad oggi oltre 300.000 imprese hanno chiuso, buttando in mezzo alla strada migliaia di lavoratori, padri e madri di famiglia che si ritroveranno da soli ad affrontare la più grave crisi lavorativa dal dopoguerra ad oggi. Ma Fratelli d'Italia sarà sempre presente e propositivo affinché si possano accogliere le proposte che presenta a vantaggio di tutte queste categorie.

si interviene con una serie di misure finalizzate ad alleggerire il peso dei costi fissi e dei costi delle imprese e delle partite IVA.

pesantemente sulle spalle delle persone. Si interviene sulla salute: è già stato ricordato nel dibattito di oggi che i vaccini e il completamento di un percorso di rafforzamento del del sistema sanitario sono probabilmente la prima e più importante misura di ripresa cui è chiamato il Paese. E poi gli enti territoriali: tutti abbiamo sperimentato quanto sia fondamentale, in momenti di criticità e di pesantezza come quella che siamo chiamati ad attraversare, avere degli enti locali (amministrazioni comunali e non soltanto) capaci di intervenire là dove ci sono le maggiori e più pesanti criticità.

di ripresa e resilienza su cui tutti facciamo affidamento per dare una prospettiva al Paese. Credo che bene si sia fatto a mettere in campo questo e il prossimo provvedimento, perché dobbiamo arrivare ad avere un tessuto sociale e un sistema imprenditoriale in grado di affrontare quel percorso di rilancio e resilienza che ci prefiggiamo di affrontare. Per quanto riguarda il comparto agricolo, che ho seguito particolarmente in questa vicenda, avevamo avuto nell'articolo 39 un incremento rilevante di risorse per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura, a cui in sede di conversione si sono aggiunti alcuni provvedimenti che credo siano molto importanti:

che permetta loro di potervi accedere; infatti il credito di imposta come sistema fiscale delle imprese agricole è in molti casi un enunciato di fatto poi non percorribile. La norma sull'utilizzabilità dei prodotti etichettati senza i requisiti UE, per le imprese che in questo anno hanno faticato ad adeguarsi da una parte e dall'altra parte in molti casi hanno i magazzini pieni di etichette, perché si è venduto molto meno, permetterà di avere più tempo per poter chiudere

entrando in pista nel nostro Paese e può garantire un'ulteriore opportunità di sviluppo importante. Non avevamo però una norma che permettesse di definire in modo puntuale come dovevano mettersi in campo queste aziende per poter commercializzare il loro prodotto. Nel decreto-legge in esame abbiamo pertanto approvato questo testo. C'è poi anche il tema degli esoneri contributivi per le aziende agricole. noi eravamo partiti con un'ambizione diversa: quella di affrontare anche molti altri temi importanti, a partire dalla risposta al problema dei lavoratori stagionali in agricoltura. Qui c'è un tema importante: il costo purtroppo esoso di questo provvedimento non ci ha permesso di risolverlo in questa sede, ma nell'ordine del giorno richiediamo con forza al Governo che, nel prossimo decreto, sia contemplata questa misura, perché una marea di persone non hanno potuto fare il minimo di giornate lavorative necessarie

di dare risposte alle problematiche della zootecnia da carne. Avevamo ipotizzato in questo provvedimento di lavorare sulla percentuale di compensazione IVA, ma anche in questo caso, per mancanza di risorse, non è stato possibile completare il percorso. il tema degli agriturismi, la norma di chiarimento sulla connessione, su cui da anni si sta lavorando, diventa elemento molto importante per dare prospettive e opportunità di crescita a questo comparto. il tema dei chiarimenti sulla dieta e l'approvvigionamento di reflui per gli impianti anaerobici per la produzione di elettricità e biometano. Sono tutti interventi che dovranno andare a sommarsi a un incremento di risorse per quel che riguarda il fondo delle filiere. Noi sappiamo che l'agricoltura - lo dicono tutti i numeri - è uno straordinario settore in termini di opportunità in generale, e soprattutto per alcuni territori marginali, nei quali la scommessa sul futuro o è agricola o non lo Perché questo possa avvenire, però, serve un rafforzamento delle filiere. Questo anno abbiamo approvato provvedimenti importanti, che vanno nella logica di innestare maggiore equità all'interno dei singoli segmenti del settore, ma è chiaro che una ristrutturazione del settore chiede risorse. Quindi, abbiamo chiesto e chiederemo un rafforzamento delle risorse nel decreto-legge che è prossimo ad emanarsi. È necessario poi un intervento a favore dei piccoli

dire che si è lavorato molto bene e credo che questo possa essere di premessa per i prossimi provvedimenti su cui il Paese confida in modo importante per poter guardare con maggiore fiducia al futuro.

Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare»

*(M5S)*. Signora Presidente, dal tentativo di censura di cui si discute da qualche giorno - mi riferisco alla ormai famosa telefonata tra Fedez, la vice direttrice di RAI 3 e soggetti legati alla produzione del concertone del primo maggio il messaggio agghiacciante che ne viene fuori, che è stato esplicitamente e più volte ripetuto durante la telefonata, è che c'è un sistema e bisogna ad esso adeguarsi. adeguarsi. Secondo i censori esiste quindi un sistema in cui un artista, in un programma che va in onda sulla RAI, non può raccontare fatti gravi, realmente avvenuti. Ripeto: fatti, non opinioni. Non può dire che un consigliere regionale leghista ha dichiarato «se avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno», oppure citare altre dichiarazioni di questo tenore omofobico. Fortunatamente il tentativo di censura non è andato a buon fine, perché Fedez si è ribellato, non si è fatto intimidire, non ha pensato a ricadute negative per la sua carriera, ma anzi ha reso pubblico quanto accaduto. Il solo fatto però che qualcuno abbia tentato di controllare le parole di un artista è di una gravità inaudita. I casi sono due: o si è trattato di un tentativo di censura spontaneo da parte della vice direttrice di RAI 3 o di chi le ha detto di intervenire in quel senso, oppure è stato un tentativo che è stato conseguente ad una precisa richiesta di una parte politica. Entrambe le ipotesi sono gravissime e non possono rimanere impunite. Chi ha sbagliato deve pagare, deve assumersi le proprie responsabilità e coloro che in RAI hanno tentato di censurare devono dimettersi immediatamente. Tra l'altro, nel caso specifico, la televisione di Stato aveva acquistato quello spettacolo confezionato al di fuori della RAI e, quindi, è ancora più difficile comprendere il motivo per cui l'azienda, oppure solo alcuni dei suoi dirigenti, erano preoccupati per uno spettacolo organizzato dai sindacati e prodotto da una ditta esterna. In questa vicenda non discutiamo di un errore o di qualcuno che è stato più realista del re: re: c'è in ballo la tutela della libertà di espressione. Non lo dico perché concordo con l'intervento di Fedez, ma per affermare un principio irrinunciabile. Tutto questo non sarebbe mai accaduto in un'azienda libera e indipendente, e se succede, è perché la RAI è lottizzata e non certo da ieri. e non certo da ieri. È nostro dovere riformare questo grande presidio culturale italiano perché tutto ciò non avvenga più e, per farlo, occorre che le forze politiche, tutte, rimangano fuori dall'azienda. Chi lavora in RAI, a qualsiasi livello, deve poterlo fare per merito, per riconosciute e dimostrabili capacità professionali e non per appartenenza politica.

«Roma: giovane lesbica rifiutata al colloquio di lavoro. "A noi servono donne, non maschi mancati"». «Cagliari: bulli aggrediscono diciassettenne omosessuale e la sua amica; il video *choc* su Facebook». «Gay picchiato dal branco a Tiburtina. "Ecco come trattiamo quelli come te a Roma"». Potrei andare avanti. Questi sono casi di cronaca, Presidente, del 2019, quando io depositai il mio disegno di legge in materia di contrasto al fenomeno dell'omotransfobia. Allora non se ne parlava, oggi per fortuna se ne parla, ma questi casi sono sempre successi e purtroppo continueranno a succedere, a meno che

Francia 2004, Germania 1992, Grecia 2005, Irlanda 1993, Islanda, Lussemburgo e Norvegia 1981, Olanda 1991, Romania 2002, Spagna 2003, Svizzera 1999. In Svezia il reato di incitamento all'odio contro le persone LGBT è stato inserito in Costituzione nel 2002 e non è cascato il mondo e la Svezia esiste ancora. Infine, nel Regno Unito esiste una legge di contrasto all'omolesbobitransfobia dal 2005. Questa legge in Italia ha avuto una gestazione lunghissima: tredici anni fa è stato fatto il primo tentativo di approvazione; poi c'è stato il grande lavoro di concertazione bicamerale messo su da Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico. Oggi Lega e Forza Italia annunciano improvvisamente che presenteranno un loro disegno di legge alternativo a quello già approvato a larga maggioranza alla Camera, dimostrando scarsa scarsa sensibilità democratica e scarso rispetto delle istituzioni, perché vogliono bypassare un testo di legge già approvato alla Camera, spericolata volontà di improvvisazione e strumentalità. Si tratta di tecniche dilatorie. Se questo tema gli fosse veramente interessato, avrebbero avuto tre anni per legiferare in materia e non c'è alcun disegno di legge di queste forze politiche. Sono ventisette anni che l'Italia aspetta questo disegno di legge. Ora basta prese in giro. Se si intende continuare così, il MoVimento 5 Stelle ha già raggiunto più del numero sufficiente ad attivare l'articolo 77 e a chiedere la calendarizzazione direttamente in Aula. Fissiamo un termine per l'Aula e dimostriamo che la nostra volontà di approvare la legge Zan contro omofobia, misoginia

Signor Presidente, è difficile accettare che anche lo Stato, che avrebbe dovuto essere uno dei pochi presidi di legalità in una Calabria abbandonata da tutti, invece nel caso delle scuole si sottragga in modo vile al proprio ruolo e alla propria funzione. Al degrado economico e produttivo del territorio si è aggiunto il fatto che la scuola facilmente sia diventata la passerella più a buon mercato per politici spregiudicati che hanno abusato e abusano del proprio ruolo istituzionale. Dal presidente facente funzioni Spirlì, che ha inaugurato la stagione delle chiusure delle scuole di ogni ordine e grado anche in zona giallo-arancione, al sindaco Alecci, arrivato a far chiudere per un giorno la classe della scuola dell'infanzia frequentata dal bambino autistico di Soverato cui la dirigente scolastica aveva rifiutato l'affiancamento in classe da parte del terapista Abba pagato dalla famiglia, ormai è diventata una prassi per gli amministratori calabresi fare prove di forza con la scuola, nella totale inerzia del Ministero. La situazione esplosiva dipende anche dagli uffici periferici del Ministero. Dopo il caso dell'arresto del dirigente dell'ufficio territoriale di Catanzaro, la sospensione della direttrice dell'ufficio scolastico regionale, si va a ripescare, per collocarlo nell'ufficio scolastico di Catanzaro, un dirigente plurisanzionato proveniente dall'ambito provinciale di Cosenza, il dottor Luciano Greco, mentre l'ambito territoriale di Cosenza rimane ancora una volta sprovvisto di dirigente. Questa situazione è indicativa del trattamento riservato alla Calabria dal Ministero: siamo considerati meno di zero. Ma non finisce qui. Ho presentato ormai da oltre un anno un'interrogazione rimasta rigorosamente senza risposta sull'operato di una dirigente scolastica di un istituto professionale di Lamezia Terme, la quale dal 2018 ad oggi avrebbe compiuto diversi atti illeciti: ha certamente cambiato il docente di diritto a ben otto classi nel mese di maggio 2018; avrebbe dirottato l'iscrizione al terzo anno degli studenti dall'indirizzo commerciale a quello alberghiero senza previa acquisizione del loro consenso; avrebbe lasciato che il proprio collaboratore operasse con diverse sovrapposizioni di più classi nelle stesse ore, abbinandolo illecitamente per un complessivo settimanale inferiore alle diciotto Tutto ciò è stato segnalato invano: gli uffici del Ministero rimangono totalmente inerti; nessuno risponde alle interrogazioni su questi fatti che mettono a nudo un sistema palesemente insostenibile. A cosa servono i dirigenti e i funzionari del Ministero se si limitano a mettere pezze o la polvere sotto al tappeto rispetto ad una gestione che è diventata un colabrodo?

Signor Presidente, questa volta possiamo sperare in un intervento concreto a favore delle infrastrutture necessarie per rivitalizzare la Sardegna centrale? Avremo il coraggio di invertire una tendenza che diversamente porterà le zone interne ad un irreversibile declino? È recente la presentazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle schede *recovery fund* per la Regione Sardegna, ad opera dell'Assessorato ai trasporti che - come tutti noi - spera in un attento e risolutivo intervento. Il primo riguarda la rete ferroviaria Nuoro-Macomer, che ha tutti i requisiti previsti: la tempistica di quattro anni e mezzo, gli oneri finanziari di 114 milioni di euro e l'impegno della Regione Sardegna a cedere la linea ferroviaria alla Rete ferroviaria italiana. Nuoro è l'unico capoluogo di provincia nazionale a non essere attraversato da un sistema ferroviario nazionale. A oggi l'accessibilità al capoluogo è garantita da soli mezzi su strada. Dalla linea nazionale vengono completamente esclusi tutta l'area vasta del centro Sardegna e l'intero versante della Sardegna orientale, ambiti che nei decenni scorsi hanno sofferto tantissimo per queste limitazioni. sarebbe l'occasione - come indicato dal ministro Giovannini - per sanare il disequilibrio, realizzando il completamento della rete ferroviaria sarda servendo i territori centrali e orientali. In questo modo garantiremo a tutto il centro dell'isola - in particolare a Nuoro - un sistema di collegamento ferroviario con i principali porti di Cagliari e Porto Torres e con l'aeroporto di Cagliari e, quindi, le connessioni con le TEN-T europee. Favoriremo inoltre la connessione veloce, sicura e *green* fra i poli produttivi dell'isola e il trasporto delle merci da Pratosardo a Bolotana, verso gli scali marittimi di Cagliari e Porto Torres. Rafforzeremo, mediante il sistema ferrato, i collegamenti tra la parte orientale e occidentale dell'isola, consolidando le attività turistiche. Sosterremo la transizione verde, supportando la mobilità sostenibile: le stazioni dovranno essere moderne, i treni agibili ai diversamente abili. Aumenteremo il potenziale di crescita economico ed occupazionale e favoriremo l'insediamento di nuove attività per contrastare lo spopolamento. Se non coglieremo queste possibilità e non ci batteremo per realizzare le infrastrutture avremo grosse responsabilità

Sarebbe un bellissimo riconoscimento aiutare a creare le condizioni per permettere alla provincia di Nuoro un progresso civile ed economico. c'è una questione che mi sta particolarmente a cuore e che ritengo doveroso far presente, poiché anche nell'emergenza che attraversiamo dobbiamo salvaguardare le iniziative meritevoli e di prospettiva. Proprio queste caratteristiche incarnano le Universiadi, una manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai Giochi olimpici, ma in ambito universitario. Il suo svolgimento è biennale e vi partecipano atleti provenienti da ogni parte del mondo. Torino si è candidata a ospitare l'edizione dell'evento nel 2025 in quanto ha già attivato tutte le procedure necessarie e sta dimostrando la volontà e il valore di tutti gli attori locali nel perseguire tale obiettivo. Lo svolgimento dei Giochi mondiali universiadi invernali 2025 comporterà un incremento di visibilità a livello nazionale e internazionale del territorio piemontese; un potenziamento dell'attrattività economica del territorio; un significativo e duraturo ammodernamento delle strutture sportive pubbliche e costituirà un volano per la promozione della cultura dello sport e della sana competizione, oltre a valorizzare il territorio come meta di nuovi visitatori. La Regione Piemonte ha già previsto all'interno del proprio bilancio uno stanziamento per il sostegno dell'evento, ma ora il Governo deve fare altrettanto, formalizzando la disponibilità delle garanzie economiche per la sua organizzazione. Il 14 maggio è la data prevista per la firma del contratto firma del contratto e manca pochissimo. Senza garanzie da parte dello Stato almeno delle risorse per l'avvio della macchina (5 milioni di euro sui 28 previsti in spesa corrente da qui al 2025),

in Senato ad un imprenditore che penso meriti da parte di tutta l'Assemblea una gratitudine autentica per un atto di autentica civiltà. L'imprenditore è Giuseppe Condorelli. *(Applausi)*. Da notizie di stampa

questo atto di coraggio che è nella scia e non rende vano il sacrificio di quanti hanno avuto il coraggio di denunciare, a partire da Libero Grassi.